essere sempre cauti nell'utilizzazione della norma penale. Dobbiamo costruirla bene, costruirla in modo tecnicamente corretto. Questa è almeno la seconda volta dall'inizio della legislatura che la norma penale viene modificata

emanare una norma penale, che naturalmente ha effetto sulle libertà personali, attraverso un decreto-legge non è una buona pratica, soprattutto da parte di un Governo che, tra l'altro suscitando la nostra grande attenzione, ha molto insistito sul tema del garantismo. Voglio anche aggiungere un altro elemento di tipo tecnico: questo è il primo caso - ma sappiamo che nell'altro ramo del Parlamento se ne sta discutendo - di un reato cosiddetto universale, cioè un reato che sarebbe imputabile alle persone che lo hanno commesso anche se lo avessero commesso fuori dal nostro Paese. Anche questo è un istituto che certamente esiste, che dev'essere applicato se necessario (in caso per esempio di genocidio, siamo tutti d'accordo che il reato debba essere universale). Non dico che nello specifico questo non sia il caso, ma ancora una volta penso che non sia materia sulla quale legiferare con un decreto-legge, perché si tratta di materia assolutamente eccezionale. Se si aggiunge che nell'altro ramo del Parlamento si sta parlando di un altro reato di tipo di tipo universale, cominciano a diventare tanti. Se si tratta di un caso eccezionale e il Parlamento italiano è occupato in tutte e due le Camere per discutere di un reato universale, c'è qualcosa che non va. Inoltre, questo reato è molto indeterminato, nel senso che a leggere la fattispecie

possano essere valutati anche dal giudice. Lasciatemi ricordare la recente sentenza della Corte costituzionale sul caso Cospito, che secondo me non è stata una sentenza politica, ma una sentenza tecnica, che se una norma prevede che il giudice non abbia la possibilità di introdurre delle attenuanti su una certa fattispecie, questo ingabbia il giudice e lo priva di una possibilità di valutare il fatto che sta scritta dentro la nostra Costituzione. Come dunque faccio in modo diuturno nella Commissione giustizia, mi sforzo ancora una volta qui in Aula di di sottolineare il nostro apprezzamento per le linee programmatiche del Governo in tema di diritto penale, che ci vedono molto favorevoli, ma richiamo il Governo e la maggioranza a una maggiore coerenza con quelle linee, perché è importante che noi sposiamo il garantismo. Come sapete, il Gruppo a nome del quale vi parlo è fortemente garantista, quindi il nostro incoraggiamento è a essere più cauti più tecnicamente prudenti, perché il rischio è di produrre norme penali mal funzionanti e dato che le norme penali incidono sulla libertà delle persone (tema che a volte passa un

che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

legge; ma, siccome c'è un'indeterminatezza della norma incriminatrice, per come l'avete voluta scrivere, evidentemente c'è bisogno di tale specifica, perché non vorremmo che costituisse una forma di intimidazione

uno di questi è la determinatezza delle condotte, quando stabiliscono una pena. Vorrei facilitarvi il compito, quindi richiamandomi a qualche riferimento culturale più facile per voi: persino il codice Rocco... almeno sotto questo punto di vista con una chiarezza espositiva di determinatezza delle condotte. di garantismo è parlare a sproposito o comunque una citazione puramente di maniera per chiedere salvacondotti per alcuni, in questo caso ben determinati.

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 10 parla della creazione dei centri di permanenza per il rimpatrio e quindi prevede che, ai fini di una rapida implementazione, per aumentare la disponibilità dei posti, si agevoli la procedura dell'individuazione delle strutture. Quindi i prefetti, che sono incaricati dell'individuazione delle strutture, possono agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, antimafia e di prevenzione. A questo punto io ho chiesto e insisto nel chiedere che vengano altresì rispettate le norme in tema di codice in materia ambientale e dei beni culturali.

alle norme ambientali e sui beni culturali, si creerebbe un danno permanente all'ambiente e ai beni culturali. Quindi, chiedo al Governo e alla maggioranza di prendere in considerazione il fatto che il prefetto, nel suo agire, tenga in considerazione anche il rispetto dell'ambiente e dei beni culturali. Diversamente gli italiani, per creare più posti per accogliere gli immigrati, distruggerebbero per sempre il proprio ambiente e i propri beni culturali. Invito pertanto la maggioranza a mutare il proprio parere. Nella denegata ipotesi in cui non se ne convincesse, chiedo che l'emendamento venga trasformato quantomeno in un ordine del giorno e conseguentemente accolto.

Quello che ci preoccupa davvero è la gestione, l'idea delle deroghe, la mancanza di una vera garanzia sui diritti delle persone che saranno trattenute in questi luoghi. Da questo punto

e sperare che da parte del Parlamento sia prestata una grande attenzione al rispetto dei diritti umani, delle condizioni igienico-sanitarie, dei diritti delle persone, dei nuclei familiari e delle persone che hanno problemi, attraverso l'assistenza necessaria.

I CIE non ci sono più e sono stati trasformati in Centri per il rimpatrio (CPR); li ha trasformati il centrosinistra

molte Regioni e le Forze di polizia su tutto il territorio nazionale. Cito come esempio la Regione Emilia Romagna, che non ha un Centro per il rimpatrio, e, quando c'è bisogno di rimpatriare qualcuno, le Forze di polizia locali devono andare in giro per l'Italia a cercare un posto.

carcerarie perché hanno commesso gravi reati sul territorio e, se non venissero espulsi immediatamente e portati in un Centro per il rimpatrio, tornerebbero a delinquere sul territorio. Questo è quello che c'è nella maggior parte dei Centri per il rimpatrio, proprio per la loro capienza molto limitata. Questa maggioranza e questo Governo intendono puntare sui rimpatri, perché è indispensabile

procedura di espulsione più veloce, perché nel territorio della nostra Nazione non ci può stare chi delinque. vorrei semplicemente dire al collega Lisei che non si deve meravigliare, perché siamo di fronte al classico caso dell'ipocrisia di chi predica la solidarietà e l'accoglienza, ma a casa degli altri.

Signor Presidente, più andiamo avanti con la legislatura e più si evidenziano le differenze che ci sono tra le varie forze politiche in campo e quelle che ci sono all'interno del Parlamento, ed è bene che questo sia: è bene che vi siano queste differenze, perché è il sale della politica. *(Brusio)*.

sul territorio nazionale e che sono rappresentate in Parlamento, ma è giusto che questo sia: è il sale della democrazia il fatto che ci sia la possibilità di confrontarsi su qualsiasi tipo di argomento e che ci siano

nel corso dei secoli hanno fatto parte dell'essere umano, della vita dell'uomo. Noi siamo stati tra i protagonisti della migrazione verso altri territori per poter crescere,

il pensiero di essere depositari del giusto e della verità, ma non è così. Noi ci sentiamo persone autorevoli, tanto da poter mettere in campo le nostre idee, i nostri pensieri e le nostre soluzioni. Le nostre sono soluzioni che reputiamo valide hanno ricevuto il consenso popolare, che ci ha permesso di portarle avanti. Lo facciamo con grande impegno, con grande voglia e con grande volontà, ma nel rispetto dell'avversario politico. L'avversario politico va rispettato. Noi reputiamo di avere

di portare avanti ciò in cui crede. Fortunatamente, rispetto agli anni passati, abbiamo un Governo politico che ha una visione e un obiettivo: su questo si deve

all'immane tragedia di Cutro del 25 e 26 febbraio. Era necessaria e urgente una risposta a quell'orrore, con 94 vittime accertate - come sappiamo

profondamente sbagliata, anche perché quell'orrore, quello del Mediterraneo, rischia di continuare ancora: continuano a morire migliaia di persone ogni anno e porre fine a quella strage è un dovere umano, civile e democratico. Ci si sarebbe aspettati almeno un guizzo di

che però è rigorosamente coerente, ad esempio, con la dichiarazione del Ministro dell'interno subito dopo il naufragio, ma anche con la scelta gravissima dello stesso presidente Meloni - non dimentichiamolo - che non volle incontrare i parenti delle vittime a Cutro, forse per non irritare una parte del proprio elettorato. Fu annunciata in quei giorni una guerra senza quartiere contro i trafficanti,

essi stessi nelle barche, a guidarle, magari con il rischio di annegare pure loro? Non vi viene in mente, ad esempio, che la realtà è invece profondamente diversa da questa narrazione propagandistica e che il timone di quelle barche venga spesso affidato proprio a qualcuno di quei disperati, che si mettono in mare a sfidare le onde? Quelli a cui volete dare la caccia, spesso, sono l'ultima ruota del carro, se non l'ultimissima; sono quelli che addirittura, a volte, non hanno nemmeno i soldi per pagarsi il viaggio e proprio per questo accettano di guidare i barconi. Della loro sorte, evidentemente, ai trafficanti non importa nulla. Aumentare le pene, come ben si vede, non risolve il problema. L'altra formula sulla quale puntate sarebbero gli accordi con i Paesi da cui partono le barche, compensati per la loro collaborazione. Come però sappiamo, sono spesso Paesi che ignorano i diritti umani si può facilmente immaginare come si adopereranno per fermare le partenze. In realtà, non c'è nemmeno particolare bisogno di usare l'immaginazione: basta guardare a quello che succede quotidianamente in Libia, alle torture, agli stupri, agli omicidi e ai *lager* che noi finanziamo. È una macchia vera e propria che l'Italia e l'Europa non riusciranno a lavare facilmente; una colpa che dovrebbe davvero farci vergognare di noi stessi e della nostra sedicente civiltà. Dovremmo chiederci fino a quando volteremo la testa dall'altra parte per non guardare. E invece vogliamo moltiplicare il modello libico o ancora l'accordo che avete trovato sulla protezione speciale. Ieri siete stati obbligati a una mezza marcia indietro, e questo naturalmente è un bene, ma l'attacco che avete fatto alla protezione speciale resta una scelta gravissima, giustificata con vere e proprie menzogne. Il presidente Meloni ha detto che questa protezione esiste solo in Italia. Non è vero: esiste in 18 Paesi europei. Dite che è un fattore di attrazione verso il nostro Paese. Non è vero: le richieste di questo tipo esempio, dalla Germania, Paese non di primo sbarco, sono state il triplo delle nostre, che sono comunque poco più di 10.000, numeri evidentemente molto diversi dalla cosiddetta invasione di cui a sproposito parlate. Il Governo giustifica questa irragionevole stretta con la necessità di fermare gli sbarchi, ma non è vero neppure questo. La grande maggioranza della protezione speciale è stata riconosciuta a immigrati dal Sud America o dai Balcani, che evidentemente non arrivano dal mare. La verità è che questa norma, come la guerra insensata che avete fatto e che state facendo alle ONG o come la stessa dichiarazione dello stato di emergenza, ha il solo scopo di creare un clima isterico e di destare un allarme sproporzionato a puri e meschini fini di propaganda. *(Applausi)*. I Comuni e le Regioni che bocciano questa linea non lo fanno per calcolo politico, ma perché sanno che essa sarà non solo inutile, ma anche dannosa, perché moltiplicherà evidentemente e ovviamente il numero degli irregolari. La stessa riapertura dei flussi sarebbe giusta se i numeri di cui si parla non fossero così insufficienti come sono e se non ci fosse naturalmente di mezzo una legge sbagliata come la Bossi-Fini. Tutti sanno, finanche chi l'ha scritta, che quella legge andrebbe cambiata. Tutti sanno, innanzitutto le imprese, che i flussi previsti sono insufficienti per la nostra economia. Tutti sanno che un crollo degli arrivi sarebbe devastante per il nostro Paese, a partire dal Governo stesso, che peraltro lo ha scritto candidamente nel DEF. Tutti sanno che i migranti potrebbero essere una risorsa e non un problema. Tutti lo sanno, tranne evidentemente quelli che vaneggiano di sostituzione etnica, com'è stato fatto in questi giorni. *(Applausi)*. Come si vede, allora, il provvedimento va anche contro gli interessi reali del Paese, oltre che contro i principi elementari di civiltà, solidarietà e umanità. Penso, lo dico al Governo - che non riuscirete a cancellare quella civiltà giuridica e politica che già nella seconda parte del Novecento seppe dare in Italia e in tutta Europa la giusta dimensione alle grandi questioni di cui stiamo parlando. Il premio Nobel Heinrich Böll scrisse che il nostro tempo, semmai avrà un nome, sarà chiamato il secolo dei rifugiati. I nostri Padri costituenti vollero scolpire quei concetti nella solennità dell'articolo 10, quello relativo al diritto d'asilo;

e, oggi, anche dei cambiamenti climatici. Non dimenticatelo. Non dimentichiamolo mai. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, dopo il terribile naufragio avvenuto tra il 25 e il 26 febbraio a poche centinaia di metri dalla costa calabra, in località Cutro, che ha causato la morte di ben 94 persone oltre a un numero imprecisato di dispersi, il Governo avrebbe dovuto avviare un confronto con tutte le forze politiche e con i soggetti che a vario titolo operano nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione, avviando un *iter* legislativo per la modifica delle disposizioni in tema di immigrazione in modo ragionato e condiviso. però non è stato, perché ancora una volta il Governo ha scelto di utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza per legiferare, impedendo al Parlamento di svolgere il proprio ruolo e spegnendo qualsiasi tentativo di confronto e di dibattito nella pervicace convinzione di avere le risposte giuste ad ogni problema. Eppure questo provvedimento, lungi dall'introdurre modifiche migliorative al testo unico sull'immigrazione, indebolisce il sistema dell'accoglienza, con il tentativo di parte della maggioranza di reintrodurre le norme del vecchio decreto Salvini, che sollevarono e continuano a sollevare

del fenomeno - come dimostra la storia di questi vent'anni, da quando cioè è stato introdotto il reato d'immigrazione clandestina - non ha sortito alcun effetto deterrente sulle partenze. Lo vediamo anche in queste settimane: dopo il decreto contro le ONG, gli arrivi sono triplicati. pericoloso, perché l'unico effetto concreto sarà quello di spingere sempre più i migranti ai margini della legalità, come hanno ben spiegato tanti amministratori locali. Ciò che serve sono politiche e strumenti d'integrazione sociale. Bisogna operare una semplificazione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno e per l'impiego degli immigrati nel tessuto economico. Quello che non serve, invece, è la cancellazione delle forme di protezione, di più gli immigrati alla mercé della criminalità organizzata, che è continuamente alla ricerca di manovalanza per le proprie attività. Allora, se un merito vogliamo riconoscere a questo provvedimento, è quello di aver reso evidente un approccio ideologico che - come ha ben spiegato ieri anche il collega Filippo Sensi - presto andrà a sbattere contro le realtà che oggi vengono negate. Mi hanno molto colpita le parole del ministro Lollobrigida, rispetto alle quali esprimo forte e chiaro il mio aperto dissenso e la mia condanna morale. No, signor Ministro, in Italia non è in atto alcuna sostituzione etnica. Trovo anzi pericoloso diffondere simili suggestioni, conferendo loro una sorta di legittimazione istituzionale. Se arriva a dichiararlo un Ministro, allora sarà vero che esiste un disegno per sostituire gli italiani con gli immigrati: è questo ciò che rischiamo di far pensare agli italiani.

che nulla apporta, in termini di dibattito politico, mentre si offendono gratuitamente le persone nella loro intimità familiare e nella loro vita privata. Anche questo non è dibattito politico. Al di là però dell'assoluta infondatezza storica della teoria della sostituzione etnica, sono proprio i dati sull'immigrazione a smentirvi. Dal 2011 ad oggi, infatti, la percentuale di stranieri in Italia è cresciuta di appena l'1,8 in secondo luogo, come non smettono di ripetere le categorie produttive, tra le quali una quota importante anche dei vostri elettori, l'Italia ha bisogno di manodopera. È questo un bisogno che altri Paesi, come la Germania, stanno risolvendo mettendo in diretto rapporto le domande di protezione con le domande di forza lavoro nelle imprese. Inoltre, anche i dati del Documento di economia e finanza del MEF dichiarano che, aumentando di un terzo l'immigrazione, il debito pubblico italiano scenderebbe di almeno trenta punti. una realtà quindi che, unita alla tragedia di Cutro, doveva spingere il Governo ad abbandonare i toni della propaganda e affrontare quelli d'interesse nazionale; a revisionare il testo unico dell'immigrazione con un approccio condiviso, tenendo conto dei dati del sistema economico e occupazionale, che, soprattutto per i lavori *low profile*, è sostenuto prevalentemente dagli immigrati; ad aprire i canali per un'immigrazione controllata, partendo dall'abolizione della legge Bossi-Fini, che ostacola la ricerca di manodopera per le imprese; ripristinare una missione di soccorso in mare, per obbligare anche l'Europa alla modifica di norme che - per citare le parole del presidente Mattarella - sono preistoriche; immaginare nuove politiche per l'immigrazione, un concetto purtroppo totalmente scomparso dal vocabolario della politica; non ultimo, a cancellare le norme contro le ONG, perché la solidarietà non può mai costituire un reato e il soccorso in mare, oltre che obbligatorio, costituisce il primo baluardo del diritto internazionale, che di certo non possiamo permetterci di infrangere. Per concludere, signor Presidente, la domanda che - per suo tramite - vorrei porre ai colleghi della maggioranza è se pensano davvero che il giudizio su questo Governo passerà da quanto si dimostreranno forti con i più deboli e con i disperati. Io penso invece che gli italiani giudicheranno questo Governo dal modo in cui riuscirà a spendere, se ci riuscirà, tutte le risorse del PNRR; dal modo in cui contrasterà il carovita, ridando potere d'acquisto alle famiglie; dal modo in cui interverrà sulla sanità pubblica e dall'impegno per sbloccare quell'ascensore sociale nemico del merito e delle nuove generazioni. Quel che è certo è che nessun Paese ha scritto il proprio futuro aggiungendo norme al codice penale. Soprattutto, a nessun Paese sono concesse scorciatoie, quando si è dentro cambiamenti epocali, che richiederebbero una politica che guardi ai prossimi anni e non ai sondaggi della prossima settimana. è questa la strategia del Governo, sappiate fin d'ora che sarà fallimentare, si infrangerà subito innanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia europea e, dal punto di vista storico, costituirà un fallimento sulla pelle dei più deboli e sul futuro del Paese, in spregio ai suoi valori di umanità e di solidarietà. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope per annunciare il nostro voto fermamente contrario a questo decreto-legge, che è nato già debole e completamente inadeguato al suo obiettivo. Cominciamo col dire che esso nasce dopo la strage di Cutro, purtroppo non la prima e temo non l'ultima che è avvenuta nel nostro Mar Mediterraneo, rispetto alla quale il nostro Paese naturalmente ha fatto una terribile figura. Il mondo ci ha guardati in quella situazione: siamo stati balbettanti e ancora oggi non capiamo esattamente quale sia

che li avrebbero qualificati come richiedenti asilo, ma non sono mai riusciti ad arrivare qui in Italia e a esercitare il diritto che l'articolo 10 della Costituzione riconosce loro, quello di avere asilo nel nostro Paese e di usufruire dei diritti democratici di cui noi fruiamo, perché la Costituzione così

sempre così capace e affidabile, ieri a un certo punto non sapeva più che cosa fare e, quando il senatore Gasparri ha detto che avrebbe riformulato il suo stesso emendamento in Aula, ha dovuto chiederci di sospendere i lavori per capire cosa fare. Il Governo non sapeva cosa fare in quel momento, ma il Governo non sa cosa fare in un senso ancora più strategico, che è quello che veramente mi

seppure non cambiassimo l'età pensionabile e non la diminuissimo, soltanto per l'invecchiamento della popolazione il costo di sanità e pensioni ci porterebbe a sforare il rapporto tra debito e PIL e a portarlo al 180 qual è l'unica cosa che dice il Governo che può interrompere questa spirale? Il flusso netto di immigrati deve aumentare di un terzo, quindi ci possono essere più immigrati che vengono a sostenere la spesa sociale e sanitaria di questo Paese. Lo dice questo Governo nel DEF. E cosa dice ora il Governo?

di un milione di lavoratori e che non ci sono lavoratori; l'ha detto il Governo in persona e - aggiungo - lo dicono le associazioni di categoria. In questi giorni a Milano c'è il salone del mobile e oggi il presidente di FederlegnoArredo ha detto che servono 15.000-18.000 nuovi lavoratori nel settore entro i prossimi anni. Qui al Senato abbiamo avuto il presidente di Confindustria Moda e il presidente della Camera nazionale della moda che hanno detto le stesse cose. Oggi lo dice anche il Governo: mancano un milione di persone. E poi lo dice incredibilmente anche il ministro Lollobrigida, famosissimo in questi giorni, che, sul «Corriere della Sera» di oggi, alla giornalista che gli chiede cosa volesse dire con quell'infelice espressione,

E aggiunge: «Un concetto chiaro, per dire che l'indirizzo del Governo è prendere atto di un drammatico decremento della natalità, che fa prevedere nei prossimi anni un abbattimento drammatico della nostra popolazione». Quindi, siamo tutti d'accordo sul fatto che abbiamo bisogno di persone che vengano a lavorare in questo Paese. E allora la domanda è: perché tenete nell'irregolarità persone che sono nel nostro Paese e già lavorano? *(Applausi)*. Per quale motivo quando si fa il *click day* mettete a disposizione 80.000 posti migranti che lavorano, che tra l'altro voi sostenete essere all'estero, ma sappiamo benissimo che sono in Italia, altrimenti quale imprenditore farebbe un contratto a un lavoratore che non conosce? Il vostro *click day* è una sanatoria mascherata, ma soltanto per un terzo dei richiedenti.

quando il ministro Lollobrigida dice al «Corriere della Sera» che stava parlando in positivo di migrazione legale il cui primo nemico è quella illegale? Come si fa a immigrare legalmente in questo Paese? Non c'è possibilità. Perché le persone non vengono in Italia a cercare lavoro regolarmente? Perché voi continuate a mantenere una legge - la Bossi-Fini che impedisce appunto di arrivare in Italia regolarmente *(Applausi)*,perché l'unica possibilità di arrivare in Italia è avere un rapporto di lavoro da un datore di lavoro che nemmeno ti conosce. Perché, se Perché, se siete nemici dell'immigrazione illegale, fate di tutto per spingere le persone nell'illegalità? Qual è l'obiettivo? È una domanda retorica, signora Presidente, perché la risposta ce l'abbiamo: perché tenere così alti l'attenzione e l'allarme sul tema migrazioni, da parte della destra sia di Governo sia di opposizione, ha dato loro la possibilità di lucrare un consenso sulle paure delle persone. *(Applausi)*. Questo è il fatto. E invece cosa dovrebbe fare una classe dirigente responsabile? Dovrebbe dire: abbiamo un fenomeno strutturale? Lo vogliamo gestire? Come si fa? Certamente sostenendo la natalità; sono fortissimamente favorevole a sostenere la natalità; non per niente, la nostra Elena Bonetti è l'autrice del Family act, che ha dato un potente segnale al Paese dicendo che un bambino che nasce non è un lieto evento soltanto per la famiglia in cui nasce, ma è un investimento per il Paese. Tuttavia, signor Sottosegretario, il problema qual è? Che se anche tutti gli italiani

anni, non prima; quindi, c'è certamente un problema di lungo periodo, ma la domanda che faccio a questo Governo è: come risolvete il problema di breve periodo? FederlegnoArredo, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, i datori di lavoro e le nostre famiglie che hanno bisogno di assistenza non possono aspettare venticinque anni per vedere gli effetti delle politiche della natalità. E infatti, i Paesi più avveduti del nostro fanno un lavoro molto intelligente di attrazione di migranti qualificati: per esempio, investono per attrarre nuclei familiari anziché singoli, perché capiscono che, insieme alla strategia di lungo periodo sulla natalità, bisogna risolvere un problema dei nostri imprenditori oggi, signor Sottosegretario. Non sottovaluto l'aspetto umanitario, ma in questo mio intervento ho voluto parlarne perché temo che voi l'aspetto sanitario non lo sentiate. Spero almeno che sentiate i motivi dell'economia, che sentiate i motivi dell'interesse nazionale e vi comportiate come una classe dirigente che si rispetti. Invece voi fomentate l'odio, fomentate la paura fate una cosa molto brutta: dite a questo Paese che il futuro non è un'opportunità, ma una minaccia. Voi state uccidendo - e questo è ancora più grave di quello che fate ai migranti - la possibilità che questo Paese pensi per se

Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, non abbiamo interesse ad alimentare polemiche e interventi nel ribattere a questa o a quella delle tante contumelie che vengono lanciate. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Le bugie e la verità: le bugie sono quelle che stiamo sentendo da parte dei vari Gruppi di sinistra. La verità è la natura del nostro provvedimento: questo decreto-legge - non starò qui a illustrarlo punto per punto - regolamenta i flussi i flussi e serve a regolare meglio l'ingresso di persone che vengono in Italia per lavorare, in base a un principio che anche nel passato esisteva e che non sempre è stato adottato. Il Governo ha previsto 82.000 persone, ma c'è chi dice che si può arrivare a 100.000: non sarà questo il problema,

Quindi, le bugie sono quelle che vengono da sinistra e le verità sono quelle che diciamo noi. Accanto a questa regolamentazione di flussi, ci sono norme che rendono più severa la gestione dei clandestini e tutto quello che di disordinato avviene nel Mediterraneo.

Non c'è stato il classico scenario, che a volte in Parlamento pure si attiva legittimamente, con il voto di fiducia, il voto unico, nessuno discute niente e nessuno conosce i contenuti nel dettaglio, perché chi sta in Commissione

Era un dubbio che poteva esserci. Allora, nelle leggi precedenti spesso si è richiamato il rispetto dei trattati internazionali e della Costituzione, cosa che è scontata e in una legge si può scrivere o non scrivere. Non è che in tutte le leggi italiane c'è scritto che bisogna rispettare la Costituzione e i trattati internazionali: è scontato. Se una legge non rispetta la Costituzione viene cassata e i trattati internazionali vincolano i Governi. Si era quindi deciso di rivedere alcuni testi: vogliamo lasciare questi riferimenti? Lasciamoli. Questo è successo non c'è stata marcia indietro, perché le norme più restrittive sui permessi speciali sono rimaste tutte, chiare e intere, all'interno di questo testo. *(Applausi)*. La maggioranza ha lavorato, com'è normale che sia, ognuno ha le sue sensibilità o priorità. Abbiamo fatto un emendamento unitario con i colleghi Lisei e Pirovano, con il lavoro della Commissione e la collaborazione del Governo, con il quale ci siamo confrontati. Sono materie molto complesse, in cui

che chiunque lo poteva invocare e ottenere di fatto una sanatoria surrettizia. Oggi, per avere il permesso speciale per ragioni sanitarie devi avere una patologia grave che non si può curare nel Paese di provenienza e allora occorre solidarietà umana, sociale e sanitaria. Se uno ha il morbillo, se lo curerà al Cairo o a Tunisi e non c'è bisogno di venire in Italia con un permesso speciale. *(Applausi)*. Se ha una patologia più grave, può farlo; gli aerei della nostra Aeronautica vanno a prendere bambini e persone in giro nel mondo e trasportano organi, quando c'è un trapianto da fare: figuriamoci se L'Italia non ha questo alto livello di civiltà. civiltà. Non dite bugie, quindi. La protezione speciale inserita sul lavoro? Vado per *flash*, perché il tempo si esaurisce. Uno su venti è andato a lavorare. Voi l'avete allargata nel 2020, ma noi abbiamo un mandato diverso dall'elettorato e restringiamo questa normativa nel 2023. Si chiama democrazia, alternanza dei Governi. *(Applausi)*. Altrimenti, ci sarebbe sempre il Governo del PD,

Noi facciamo sintesi e ascoltiamo il Parlamento: questo è avvenuto ieri. Non siamo degli arroganti, fiducia e museruola, come hanno fatto i Governi Conte e i Governi di altri, perché poi la democrazia la si invoca qualche volta. Abbiamo vissuto in un vero e proprio regime, senza alcun dialogo, ai tempi dei Governi Conte. Noi invece in Parlamento sappiamo seguire la logica del confronto. Per quanto riguarda i flussi, il Governo sta agendo in maniera molto ampia. Riguardo a Cutro, ieri tutti ci siamo commossi a sentire i nomi delle vittime, ma leggetevi gli esiti delle indagini della magistratura: gli assassini non sono i membri del Governo italiano, ma gli scafisti che hanno gestito in maniera turpe quei viaggi

non ho qui i nomi, altrimenti leggerei quelli degli scafisti di Cutro per tenere il Parlamento nell'indignazione. Quella è la disumanità, non un Paese che ha il 10 per cento di popolazione straniera e che apre ad altre 80.000-100.000 persone.

per aiutare gli sventurati. Le Regioni e i Comuni che rifiutano questo stato d'emergenza sono disumani: loro sono i disumani? *(Applausi)*. Come li sfamano poi? Se non hanno i soldi - e non ce li hanno - lo Stato interviene. Questo è lo stato d'emergenza. Quindi chi è che dice le bugie? Sempre gli stessi. Ricordo sempre, in questi interventi, che nel 2011 un senatore disse che c'era una guerra sbagliata. Quel senatore - che si chiama Silvio Berlusconi - disse che con la Libia bisognava negoziare,

e nella Libia? O sono quelli del centrodestra e Silvio Berlusconi i pacifisti? *(Applausi)*. Quindi non siete nemmeno i veri depositari dell'amore per la pace. A Tunisi, in questi giorni, anche il vice presidente del Consiglio Tajani ha detto di dare aiuti. Voglio dire da quest'Aula al commissario per l'economia Gentiloni (del PD, ma commissario europeo), che è andato a Tunisi anche lui e ha fatto una lista di riforme e di cose che chissà quando le farà la Tunisia: l'Europa aiuti la Tunisia, sennò per colpa di Gentiloni avremo avremo i fondamentalisti e i tagliagole a Tunisi. *(Applausi)*. Caro Gentiloni, cara Commissione europea, aiuta la Tunisia, perché la Turchia è stata aiutata, con sei miliardi, per bloccare l'emergenza siriana. Ora, siccome interessa l'Italia, l'Europa lesina. Faccio nomi e cognomi: Paolo Gentiloni. È andato lì: apra i cordoni della borsa, come ha chiesto il Governo italiano, come ha chiesto la Meloni, come hanno chiesto Tajani e tanti altri. Sennò, quando ci saranno poi quelli della *jihad* islamica, dove li mandiamo? Da Gentiloni? Non credo, ovviamente. Ecco, il piano per l'Africa, il piano Mattei: la politica che noi facciamo è quella di cui ha parlato anche il Santo Padre. Una volta, tornando da un viaggio all'estero, disse: quanti ne possiamo accogliere? Un numero limitato. E disse una frase semplice: di più non posso. Ecco, la nostra linea è quella espressa anche da Papa Francesco: di più non posso. Quanto è di più? Datevi una regolata; mi pare che siamo ben oltre il di più in Italia, anche in questi questi giorni e in questi mesi. Quindi noi siamo per il rispetto delle persone e non prendiamo lezioni da chi è favorevole all'utero in affitto e considera le donne del Terzo mondo una specie di oggetto per sfornare bambini da comprare. *(Applausi)*. Noi quelle persone le rispettiamo anche in questo: non le consideriamo persone in cui impiantare un ovulo, che casomai viene da un Paese, in un corpo più robusto di un altro Paese. Quello è razzismo, quella è una

speciale. Non abbiamo fatto nessuna retromarcia: noi andiamo avanti, ma con intelligenza, con umanità e con il rispetto del Parlamento. Per questo il Gruppo Forza Italia voterà a favore del decreto-legge

ma fin dall'inizio. Appena insediati, al grido di «pronti» in campagna elettorale, da quei grandi statisti che sono, hanno immediatamente messo a fuoco il grande problema dell'Italia, i *rave party,* emanato un decreto-legge urgente per arginare questo fenomeno che flagella il nostro Paese da Nord a Sud, con raduni molesti di giovani in tutta Italia. Avercene di giovani in giro in Italia! I giovani, invece, dall'Italia di Meloni scappano, perché non c'è futuro per i giovani nell'Italia di Meloni, altro che *rave party*. Più che pronta, la *Premier* a noi sembra disorientata e affannata. È completamente inerte su alcuni *dossier* veramente scottanti, come quelli del carovita e dei mutui alle stelle, che, quelli sì, stanno mettendo in ginocchio milioni di italiani; è inerte sulle condizioni dei lavoratori e sui salari da fame

ci hanno perforato i timpani urlando i loro *slogan*: blocchi navali, controllo delle frontiere, rimpatri forzati. Poi arriva l'incarico di Governo, gli sbarchi quadruplicano e il duo Meloni-Salvini non sa più che pesci prendere, così inizia a varare misure raffazzonate e buone solo a fare titoli di giornale, senza soluzioni reali: reali: prima il decreto-legge contro le ONG, con il divieto di salvataggi multipli (e no, hai già salvato questi, mica puoi salvare anche questi altri: mi sembra molto ragionevole). le disposizioni con cui le navi vengono mandate in giro per ore, alla ricerca di altri litorali, aggravando quindi il costo di tutta l'operazione. Anche in questo caso non ci sono soluzioni, perché il grosso degli arrivi in Italia non avviene per mare o tramite le ONG. Vi è però qualcosa che purtroppo avviene anche troppo frequentemente per mare: sto parlando delle tragedie. A volte accadono anche a poche decine di metri dalla riva, com'è successo a Steccato di Cutro. La tragica beffa abbiamo assistito attoniti alle dichiarazioni sconcertanti del ministro dell'interno Piantedosi che incolpava i morti di essere morti; abbiamo guardato increduli ad una Presidente del Consiglio che in conferenza stampa inanellava strafalcioni sulla ricostruzione dei fatti e allo stesso tempo ignorava i parenti delle vittime, mentre l'Italia oggi aspetta ancora che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini spieghi finalmente

perché affrontavamo una pandemia (se qualcuno non se lo ricordasse, significa un'epidemia di proporzioni globali), oggi usa lo stato d'emergenza per fronteggiare una situazione strutturale, come il fenomeno migratorio. Paradossi meloniani,

La modalità con cui lo avete gestito è la cifra distintiva di questa maggioranza e si può riassumere in tre caratteristiche di fondo: dilettantismo, arroganza e spaccature interne. Dilettantismo perché nella gestione di questioni strutturali non riuscite a far altro che improvvisare; arroganza perché avete ricattato il Parlamento. Vi vantate di non aver messo la fiducia, ma potete farlo solo perché le persone lì fuori non conoscono giustamente le procedure parlamentari e non possono sapere che quello che avete fatto è molto peggio che mettere la fiducia. Inviare nottetempo, la notte prima dell'approdo in Aula, un subemendamento interamente sostitutivo e diverso dal decreto originario, aggirando le regole e minacciando il Parlamento di non poter esercitare le sue prerogative, ossia emendare, significa non avere alcun rispetto delle istituzioni e quindi della democrazia. *(Applausi)*. È di una tale furbesca ignoranza, che persino voi a un certo punto ve ne siete vergognati e lo avete ritirato, ma il ricatto fatto al Parlamento resta un'onta sulla vostra etica politica, su cui avrò modo di tornare più tardi. Il decreto ha fatto emergere oltre ogni ragionevole dubbio le vostre spaccature interne: il braccio di ferro non lo avete ingaggiato solo con le opposizioni, ma tra di voi. Sulla questione della protezione speciale avete messo su un tragicomico balletto di avanzate e retromarce cui il Paese e la stampa hanno assistito attoniti. I giornalisti mi chiamavano e mi chiedevano: l'hanno tolta? Ma allora l'hanno rimessa? Ma allora l'hanno ridimensionata? Ma allora cosa fanno?». Chi lo sa? Non sapete neanche voi che cosa fare, questa è la verità. Non lo sapete perché avete mentito per decenni, dicendo che la protezione speciale esiste solo in Italia e che è un fattore di attrazione incredibile per gli stranieri - non dico *pull factor* per non beccarmi la multa da parte di Rampelli - alimentando

albanese e peruviana, che notoriamente vengono in barca in Italia, sbarcando naturalmente sulle nostre coste. Viene fuori anche che sistemi di protezione simili al nostro esistono in ben 18 Paesi europei, quindi altro che fattore di attrazione, altro che situazione anomala è quella dell'Italia. Menzogne, come sempre. Voi però insistete, perché ormai dovete tenere il punto e così l'unico risultato che otterrete alla conversione di questo decreto-legge sarà avere 10.000 irregolari in più: persone che oggi lavorano e che sono da anni nel nostro Paese si troveranno all'improvviso senza permesso, ma non potranno essere rispedite al Paese loro, come dite voi, mentendo anche in questo caso. Avranno davanti due opzioni: continuare a lavorare, ma in nero, quindi smettendo di contribuire all'erario statale, oppure finire nelle maglie della criminalità, alimentando - questa sì - l'insicurezza. Geni, geni e in malafede *(Applausi)*, perché voi queste cose le sapete benissimo. Lo sapete così bene che è legittimo chiedersi se, oltre al totale dilettantismo del Governo, non vi sia dietro anche una diabolica strategia per cui si voglia appositamente esasperare la situazione per spianare la strada ad altri provvedimenti ancora più iniqui, repressivi e disumani con cui soffiare sulle vele della vostra propaganda. Di assaggi in questo senso ne abbiamo già avuti in abbondanza e non bastano le scuse del ministro Lollobrigida circa la sostituzione etnica. infatti voi siete al Governo e siete tenuti all'obbligo della responsabilità di sapere che cosa dite e quali significati hanno le parole che pronunciate.

Fate sapere ai vostri elettori l'imbarazzo e il vicolo cieco in cui vi siete cacciati e in cui avete cacciato l'Italia. Fate sapere che in queste ore il Parlamento europeo sta discutendo di una riforma della gestione migratoria. Il MoVimento 5 Stelle fin dalla sua nascita dice che il trattato di Dublino va cambiato e lo avete siglato voi *(Applausi)*, lo hanno siglato le forze di centrodestra nel 2003.

sull'etica politica dimostrata, sullo scippo della legge Saman, sul comportamento scorrettissimo del senatore Gasparri, ma mi avvio alla conclusione. Il decreto-legge che vi accingete ad approvare è dannoso e utile solo alla vostra propaganda e non potete arrabbiarvi se qualcuno lo definisce razzista, perché sono le vostre parole e le vostre azioni a definirlo così, nessun altro: non avete altri che voi con cui prendervela. Pertanto, annuncio il voto convintamente contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

e oggi dà lezioni a noi sulla coerenza. *(Applausi)*. Coerentemente, quei decreti li abbiamo votati e quelle politiche le abbiamo affrontate, il nostro *leader* ne paga le conseguenze nei tribunali e le condividiamo anche oggi, per come sono contenute nell'attuale decreto-legge. Noi siamo coerenti, qualcun altro è trasformista. La Lega voterà a favore del decreto-legge in esame, per un motivo molto semplice: a differenza della sinistra, per noi esiste un'emergenza immigrazione,

quella che diventerà una situazione potenzialmente ingestibile per i nostri territori, per le nostre comunità e per i nostri sindaci. in questo decreto-legge diciamo sì ai flussi regolari, ai corridoi umanitari, alle procedure più snelle e veloci per l'ingresso degli stagionali impegnati in agricoltura. Diciamo sì, però, anche a pene più severe per chi è responsabile della tratta degli esseri umani. *(Applausi)*. Al di là delle strumentalizzazioni della sinistra, a Cutro è avvenuta una tragedia una tragedia che ha lasciato tutti noi nel totale sconforto, per il dramma accaduto non per responsabilità della il dramma accaduto non per responsabilità della Guardia costiera, né tantomeno del Governo o dello Stato italiani. Quella tragedia è legata al comportamento di trafficanti di uomini e di scafisti senza scrupoli, che fanno quell'attività esclusivamente per un obiettivo, ovvero per scopo di lucro, non certamente per motivi umanitari. *(Applausi)*. Quelli sono i colpevoli, non certo lo Stato italiano, il Governo e la Guardia costiera! diciamo sì anche a strumenti più efficaci per le espulsioni, attraverso il rafforzamento delle attività dei CPR dei CPR e diciamo chiaramente no all'utilizzo della protezione speciale come una sanatoria indiscriminata. *(Applausi)*. Questi sono i contenuti del decreto-legge sui quali la Lega voterà a favore. Gli esponenti della sinistra hanno dichiarato, in questo dibattito, che i numeri attuali dell'immigrazione non rappresentano un'emergenza. Noi non la pensiamo allo stesso modo,

e 2016, in cui c'erano Governi di sinistra, nei quali abbiamo assistito al *business* delle cooperative, alle tendopoli, all'arrivo nei Comuni, senza preavviso nei confronti dei sindaci, di *pullman* carichi di migranti. Quella, sì, è stata una gestione irresponsabile che ha scaricato sul territorio l'emergenza. Di fronte all'emergenza attuale, che noi riconosciamo, non ci sono responsabilità dirette di questo Governo o dell'Italia. Non è il Governo italiano che incentiva le partenze, come venne fatto allora con lo strumento di Mare nostrum, gestito dalla sinistra. Ci sono fattori contingenti che hanno fatto impennare i numeri degli arrivi. Si tratta di fattori internazionali e di instabilità regionali che sono sotto gli occhi di tutti: il conflitto in Ucraina e quindi profughi da quel territorio e gli aumenti del costo dell'energia, cui si è accompagnato un aumento dei prezzi dei beni alimentari, che è un fattore esplosivo in Africa e che ha fatto aumentare ancora di più le partenze. C'è una grave crisi in Tunisia che è sotto gli occhi di tutti; una difficoltà di natura economica e finanziaria. Abbiamo ascoltato le parole del presidente Saïed che ha invitato i migranti subsahariani, che attualmente sono occupati, lavorano e vivono in quel territorio, a lasciare la Tunisia. Abbiamo la consueta instabilità libica. Abbiamo una rotta balcanica che ha preso la direzione del mare verso la Calabria dall'Afghanistan e dall'Iran. La somma di tutte queste situazioni sta diventando esplosiva per il nostro territorio

tema della protezione speciale. Primo punto: nessuno si può permettere di insegnare o dare lezioni all'Italia sul tema dell'accoglienza, al di là dei Governi che si sono succeduti. l'Italia ha nella propria cultura il rispetto della dignità umana come principio fondante della propria identità. Non è un tema che divide la destra o la sinistra, ma appartiene all'indole del nostro popolo. Nessun Paese europeo si sta facendo carico oggi, come nel passato, dei costi e del peso dell'accoglienza quanto l'Italia; quindi nessuna lezione, da nessuno, tanto meno dalla sinistra italiana. La protezione speciale - va chiarito - continuerà ad essere garantita. Sul tema c'è stata molta propaganda da parte della sinistra, in Commissione e in Aula. Vorrei chiarire a tutti, anche se non dovrebbe essere necessario, che per chi è oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politica, chi rischia di essere sottoposto a torture, per i minori non accompagnati o per chi versa in gravi condizioni di salute, la protezione speciale rimarrà, così com'era garantita attraverso i decreti Salvini. Cosa cambia? Ci sono modifiche che riguardano esclusivamente gli aspetti inseriti dal Governo giallorosso, dal Governo Conte II e dal ministro Lamorgese, che estendeva questi requisiti aggiungendone anche altri, molto vaghi e di dubbia interpretazione, che venivano definiti violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del migrante. Cosa significa? Può voler dire tutto e niente. Stranieri che hanno difficili condizioni psicofisiche? Questi erano strumenti che allargavano a dismisura la possibilità di utilizzare lo strumento della protezione speciale e che l'hanno resa una sanatoria di fatto. quindi una stretta sulla protezione speciale? Sì, attraverso questo decreto-legge la stretta c'è, ma in modo assolutamente responsabile da parte di questo Governo e di questa maggioranza. Non siamo d'accordo infatti sul promuovere provvedimenti che siano assimilabili a sanatorie indiscriminate. Questi sono i dati di fatto. Quindi siamo noi a dire alla sinistra basta propaganda, basta fare propaganda. Noi diciamo alle opposizioni basta creare un clima di diffidenza verso l'Italia a livello internazionale, come se le misure varate da questo Governo fossero razziste e disumane. Così non è. Vorrei toccare un ultimo tema. Questi decreti sono sufficienti a risolvere l'emergenza immigrazione? La nostra risposta è no, non bastano, evidentemente. Il Governo italiano, qualsiasi Governo, di qualsiasi colore, può varare le leggi migliori possibili per affrontare la gestione, l'accoglienza anche la repressione e la lotta all'immigrazione clandestina, come noi riteniamo di fare attraverso questo decreto, ma da solo non ce la può fare. Chi ha gravi responsabilità non è l'Italia, ma l'Europa, ancora una volta, perché è totalmente assente.

e l'Italia è abbandonata a se stessa. Signor Presidente, in definitiva la Lega si ritiene soddisfatta per i contenuti di questo decreto-legge e per le modifiche apportate attraverso emendamenti proposti dal Governo, dalla maggioranza e dal nostro Gruppo parlamentare.

giovedì 9 marzo scorso il Consiglio dei ministri, anziché a Palazzo Chigi, si è riunito presso l'aula consiliare del Comune di Cutro. In tale sede, a pochi giorni dalla tragedia che si è consumata sulle coste della medesima cittadina, ha adottato il decreto-legge che oggi quest'Assemblea è chiamata a convertire in legge.

naufragi con morti e sofferenze come quelli avvenuti pochi giorni prima della sua adozione, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Ci saremmo aspettati che il Governo intervenisse, ad esempio, sulle modalità e sulle condizioni dell'intervento della Guardia costiera, specie quando vi è notizia di un'imbarcazione nelle vicinanze e quando la Guardia di finanza è costretta a rientrare in porto per il peggiorare delle condizioni del mare. Ci saremmo anche aspettati qualche norma in grado di dare seguito alle parole del ministro Piantedosi, con le quali promise un pronto intervento nei luoghi dai quali i migranti partono. che abbiamo ancora tutti memoria, insieme al maldestro e comunque vergognoso tentativo di attribuire la colpa dei morti in mare alle stesse vittime, dell'invito fatto dal Ministro a chi fugge da guerra, persecuzioni e carestie a non partire e attendere, perché, come disse, "vi veniamo a prendere noi". Ci saremmo dunque attesi qualche precisazione su chi sarebbe andato a prenderli e in quali luoghi e con quali mezzi li avrebbe condotti in Italia. Non abbiamo però trovato nulla di tutto ciò: nulla per garantire un più coordinato ed efficace intervento di soccorso; nulla per provare a rimuovere le cause di viaggi pericolosi, in condizioni inumane e degradanti; e non abbiamo trovato nulla di serio e adeguato per affrontare il problema, che pure nel titolo si annuncia di voler affrontare, della carenza di lavoratori nel nostro Paese, anche e soprattutto in conseguenza del calo demografico. Questo è un problema molto serio, che coinvolge il nostro intero sistema produttivo, dal settore manifatturiero a quello agroalimentare a quello turistico, senza dimenticare naturalmente quello dei servizi alla persona. Le richieste di assunzione di lavoratori non appartenenti all'Unione europea presentate dai datori di lavoro nel cosiddetto *click day* sono state oltre 240.000, più del triplo della quota prevista dal Governo. E dell'impatto positivo che l'immigrazione può avere sul nostro sistema economico il Governo, peraltro, sembra essere a conoscenza. In una nota di accompagnamento al DEF viene infatti evidenziato come il nostro debito pubblico nei prossimi quarant'anni, se la situazione rimanesse com'è ora, crescerebbe di circa una decina di punti; se l'immigrazione dovesse diminuire di un terzo, il rapporto debito-PIL salirebbe dal 144 al 220 cento; se l'immigrazione aumentasse di un terzo, quel rapporto scenderebbe invece dal 144 al 133 Anche il nostro sistema previdenziale, per rimanere in equilibrio - com'è noto - ha bisogno che il numero degli occupati non diminuisca, ma al contrario cresca e si consolidi. La situazione in cui versa il nostro sistema economico e produttivo è dunque nota, così come la crescente domanda di servizi di cura e di assistenza connessa al progressivo invecchiamento della popolazione. Eppure, nel decreto non abbiamo trovato alcuna disposizione conseguente. In compenso, abbiamo trovato un'incomprensibile restrizione della protezione speciale e in particolare l'abrogazione della protezione speciale per i casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Quale sia la ragione di una simile scelta, onorevoli colleghi, è davvero difficile capire. Al di là dei pur evidenti dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 8 della CEDU, con l'articolo 7 della Carta di Nizza e, prima ancora, con l'articolo 10 della nostra Costituzione, risulta difficile comprendere quale sarebbe il vantaggio per il nostro Paese e per i nostri concittadini di abrogare tale forma di protezione speciale. L'unico effetto di questa scelta improvvida sarà aumentare il numero di presenze irregolari e, al contempo, il contenzioso. Vorrei sommessamente ricordare al senatore Tosato che la formula "vita privata e familiare" non è priva di significato, ma è esattamente l'articolo 8 della Carta europea dei diritti dell'uomo.

contribuirà a dare luogo a una situazione che, lungi dall'essere di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare - come recita il titolo del decreto-legge finirà per alimentare lo sfruttamento e il lavoro nero e per accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità,

Voglio qui ricordare una ricerca svolta da due giovani studiosi, Luca Rondi e Lorenzo Figoni, sull'uso di psicofarmaci nei CPR, presentata nei giorni scorsi alla Camera e pubblicata sull'ultimo numero di «Altreconomia». La ricerca evidenzia una situazione preoccupante, che ci sollecita ad approfondire e a verificare con scrupolo - come abbiamo chiesto in molti emendamenti - che i fondamentali diritti umani, a partire da quello alla salute fisica e psichica, siano comunque garantiti a ogni persona. Non meno irragionevoli e lesive di basilari principi costituzionali sono le disposizioni volte a semplificare e ad accelerare l'esame delle domande e, in particolare, le procedure dell'eventuale tutela giurisdizionale. Più di un dubbio di legittimità sollevano anche le disposizioni che introducono nuove fattispecie di reato, punite con estrema severità, nei confronti di chi dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel terrario dello Stato; ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, quando dal fatto derivino - quale conseguenza non voluta - la morte di una o più persone o comunque lesioni gravi o gravissime a una o più persone, senza esplicitare - come invece abbiamo proposto di fare con più di un emendamento che non costituiscono e non possono mai costituire reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria. Onorevoli colleghi, in occasione dell'approvazione dei cosiddetti decreti Salvini e del recente decreto-legge contro le ONG, ho ricordato alcune parole di Primo Levi, che voglio anche oggi rileggere: «A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno inconsapevolmente, che "ogni straniero è nemico". Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al temine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue le conseguenze ci minacciano». Sono parole straordinarie per la loro chiarezza e terribili per il loro contenuto. Sono parole che sollecitano alla prudenza, alla necessità di mitigare e ricondurre a ragionevolezza le paure e le pulsioni all'intolleranza che albergano in ciascun essere umano; parole di saggezza e di umanità, che il Governo, ostaggio della propria demagogia, credo abbia nuovamente trascurato. Per queste ragioni vi diciamo: fermatevi! Ieri qualche segnale di resipiscenza, riscrivendo l'emendamento a prima firma Gasparri, lo avete dato. Siate conseguenti, ritirate l'intero decreto-legge. Avviamo un confronto pubblico vero, aperto, coinvolgendo gli amministratori locali e facendo tesoro delle loro competenze e delle loro esperienze, nonché dei molti che operano nonché dei molti che operano nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione, nell'interesse del Paese, della legalità e di una convivenza rispettosa dei principi costituzionali e del diritto internazionale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte.

colleghi senatori, vi confesso che, nonostante abbia parecchi anni di anzianità parlamentare, ci sono momenti - come questo

qui attorno un'aria avvelenata, ma non solo e non tanto perché apro i giornali questa mattina e vedo la disgustosa e volgare vignetta sul «Fatto Quotidiano» non soltanto perché ieri, come tutto questo ramo del Parlamento, mi sono alzato di fronte alla lettura dei quasi 100 nomi dei naufraghi di Cutro,

sul naufragio di Cutro, abbia usato quello sciacallaggio così brutto anche contro la nostra Guardia costiera e contro la nostra Guardia di finanza Come se qualcuno si compiacesse che quei cento morti in fin dei conti fossero da mettere sulla gobba della Meloni: non si fa così, è brutto. Da giorni ci state ripetendo, in questa bipartizione insopportabile, di là ci sono gli umani e di qua invece gli antiumani, là i profeti della solidarietà e qui quelli privi d'anima, lì ci sono i buoni e qui ci sono i cattivi: non si fa così, perché è giusto anche dividersi, ma bisogna rispettarsi e non si fa con la presunzione, tra l'altro, e la saccenteria per cui qualcuno ritiene di avere una sorta di primazia morale. Non è così. Allora lasciateci dire quello che è giusto dire e proviamo a ragionare di tutto questo. Noi stiamo esaminando una problematica drammaticamente complessa. Come si è aperto questo millennio? Questo è il millennio delle grandi migrazioni. È vero, e mi direte che le migrazioni esistono

per cento che resta e la stessa redistribuzione all'interno è dannatamente ingiusta. Lo sappiamo. Noi che siamo latini conosciamo bene il valore della solidarietà e della *pietas*

sempre maggiore e che prima di tutto viene intercettata da noi, perché stiamo qui. Si tratta di un'ondata confusa, in cui si mischiano soggetti che fuggono da situazioni di guerra e cercano asilo - ed è vero, ma diciamo la verità:

Oggi il mondo è cambiato anche perché le comunicazioni, la conoscenza e l'interdipendenza fanno sì che misteriosamente - ed è drammatico e ridicolo allo stesso tempo - quando arriva il profugo o il naufrago, lo si trova con il telefonino.

Allora, ho il diritto di chiedervi e di chiedere a questo Parlamento di ragionare su alcune cose: come si conciliano i nostri doveri di solidarietà con il nostro diritto e dovere di governare, per quanto è possibile, i moti migratori? Come si fanno a difendere il nostro territorio, la nostra identità, le nostre frontiere, il nostro ordine e la nostra sicurezza? Volete dire che non esistono questi fatti? Esistono, drammaticamente. Posso darvi alcuni numeri, poi direte che sbaglio? Benissimo.

oggi abbiamo un'accoglienza di circa 115.000 persone - saranno 400.000. Benissimo. Curiosamente questo dato di 400.000 corrisponde a un altro dato, che mi preoccupa drammaticamente, quello dei nati in Italia. Voi saprete forse, sulla base dei dati che ha comunicato l'Istat il 7 aprile scorso - se non sbaglio abbiamo toccato il punto *record* minimo delle nascite in Italia dall'Unità d'Italia in poi. Nel 1861, quando l'Italia aveva meno della metà dell'attuale popolazione, nascevano più italiani di quanti non ne nascano oggi (393.000). Sappiamo che i dati e le proiezioni ci dicono che questo Paese si sta drammaticamente inaridendo e che alla fine del secolo avrà probabilmente la metà degli attuali abitanti. Nel frattempo, sappiamo di avere sei milioni di cittadini italiani fuori dai confini e sei milioni di stranieri dentro i confini. Sappiamo che esiste una nuova emigrazione italiana di ragazzi che facciamo studiare nelle nostre università e che poi scappano via, perché li pagano quattro lire e preferiscono andare in Canada o in America.

di uomini e donne che arrivano dal Terzo e dal Quarto mondo. Tutto giusto. Abbiamo un dovere di solidarietà, che conosciamo, ma abbiamo anche un dovere di difesa dell'entità e dell'identità nazionale. È sbagliato dirlo? Ve lo chiedo retoricamente. Io credo di no, credo che sia giusto. È giusto chiedersi cosa sarà l'Italia tra trent'anni, tra cinquant'anni e tra cento anni? Io credo di sì. Diciamoci la verità, in breve. Ci sono due visioni ideali, politiche e filosofiche.

senza una regola determina quel che determina: nel nome di una solidarietà di questo tipo, alla fine vediamo troppi uomini che finiscono magari in fondo al mare, nel fango dello sfruttamento o nel ghetto di una periferia. Non le vedete le periferie disastrate delle nostre città?

emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare. Volete dire che è sbagliato? San Giovanni Paolo II diceva che il diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria Patria e diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione. Si può anche pensare che l'immigrazione si contrasti garantendo questo diritto primario a vivere nella propria terra e non promettendo un Eldorado che non c'è, non consentendo le tragedie del mare, non consentendo le tragedie dello sfruttamento, non consentendo quello che vediamo, giorno dopo giorno. È questo che ci hanno chiesto gli italiani. Questo è un modo evidentemente anche diverso.

Avete polemizzato sull'emergenza, se esiste o non esiste. Certo, è enorme tutto quello che accade. Oggi c'è un'emergenza, perché aver perché aver quadruplicato le presenze determina un'emergenza. Quindi il commissario all'emergenza cosa deve fare? Deve assumere misure in deroga che consentano l'apertura dei Centri di accoglienza, che consentano alla Croce rossa di operare, il potenziamento dei CPR, eccetera.

Noi abbiamo il diritto e il dovere di essere solidali, ma anche di difendere queste identità. Vi lascio con questo pensiero di Goethe: se davvero vuoi l'eredità dei tuoi padri, devi prima di tutto riconquistartela. Senatore Menia, non l'ho interrotta, ma le ho dato più tempo di quanto abbia comunque concesso anche agli altri.

di date nelle quali si fondano la convivenza civile e la democrazia dell'Italia. Sono tante le occasioni che il calendario ci offre, che noi celebriamo con sincera partecipazione, ma non crediamo che possano esserci dubbi sul fatto che il 25 aprile (Festa della liberazione), il 1° maggio (Festa del lavoro), e il 2 giugno (Festa della Repubblica) siano quelle che più di tutte costituiscono l'identità nazionale, il ponte tra memoria e futuro, il DNA, l'autobiografia di un Paese, di una Nazione, di una Patria, come la chiamavano i partigiani che andavano a rischiare la vita e anche a morire. *(Brusio).* PRESIDENTE. Chi non è interessato è pregato di lasciare l'Aula; altrimenti, deve consentire

partigiani comunisti, socialisti, cattolici popolari, azionisti, repubblicani, liberali, monarchici e militari. Pensiamo agli internati militari italiani, che furono rinchiusi in quei campi perché si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò.

regime del colonialismo, delle leggi razziali, dei rastrellamenti degli ebrei destinati a morire nei campi di concentramento, come ad Auschwitz e Birkenau, dove fu deportata anche la senatrice a vita Liliana Segre e dove proprio l'altro ieri il nostro Presidente della Repubblica ha pronunciato parole inequivocabili, dicendo che i regimi fascisti furono complici dei sanguinari carnefici nazisti. Del resto, già nel 2003 fu un importante esponente della destra come Gianfranco Fini, in visita a Gerusalemme, a parlare del fascismo come male assoluto. E proprio pochi minuti fa

a ribadire giudizi drasticamente inequivocabili su tragedie della storia del Novecento come i *lager* sovietici o i massacri staliniani. Rendiamo omaggio ogni anno alle persone massacrate nelle foibe e ai profughi giuliano-dalmati - la collega Beatrice Lorenzin lo sa - e continueremo a farlo, ma nel nostro Paese, in Italia, c'è stato un regime fascista. I comunisti italiani hanno avuto nella nostra storia doppiezze e contraddizioni, sì, ma si sono battuti per la libertà. Uno di loro, Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea costituente, ha apposto la sua firma alla Costituzione insieme a a quella del presidente De Nicola e del capo del Governo di allora, Alcide De Gasperi. E se oggi tutti noi siamo e sediamo qui, è perché in Italia ci sono stati la Resistenza e il 25 aprile.

di cui faceva parte anche Carlo Azeglio Ciampi, e pronunciò un discorso di unità nazionale che parlava di antifascismo, Costituzione e 25 aprile. Infine, signor Presidente, ricordo un episodio molto noto, che tutti abbiamo citato e citeremo e che rende bene l'idea. Vittorio Foa era un azionista, è stato un grande dirigente sindacale ed è stato nove anni in carcere a Regina Coeli. Giorgio Pisanò, invece, era un repubblichino che aveva aderito e partecipava alla Repubblica di Salò. Un giorno, dopo la guerra,

porse la mano, ma gli disse: «Caro Pisanò, oggi tu sei in Senato, ma sei in Senato perché ha vinto la mia parte. Se avesse vinto la tua in Italia, io sarei ancora in carcere». Ecco, in questo episodio c'è tutto possiamo lavorare tutti insieme, come abbiamo cercato di fare la scorsa settimana, per rimuovere l'odio degli anni Settanta, cosa diversa dal fascismo, dal regime fascista e dalle guerre, contro gli odi di oggi, i razzismi e gli antisemitismi, ma lo possiamo fare proprio perché in Italia

...più aderenti al nostro passato, ma, soprattutto, costruiremo un futuro di pace, libertà e democrazia. facoltà di parlare il senatore Speranzon per illustrare la mozione n. 44. e il fondamento di una coscienza nazionale, che vorremmo condivisa: una coscienza nazionale che abbraccia i valori della libertà, della democrazia e delle istituzioni repubblicane, che ripudia e deve ripudiare ogni forma di totalitarismo, totalitarismo, di oppressione e intolleranza. Tra le date che più hanno segnato il percorso della nostra Nazione verso l'unità, la libertà e la democrazia, ce ne sono alcune in particolare che ci terrei a elencare: il 25 aprile, Festa della liberazione; il 1° maggio, Festa del lavoro; il 2 giugno, nascita della Repubblica ed elezione dell'Assemblea costituente; il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia; il 4 novembre, Festa dell'unità d'Italia e delle Forze armate e altre importanti date che dobbiamo tenere a memoria, perché rappresentano pagine significative per la nostra comunità nazionale. Cito ad esempio quella del 27 gennaio, la Giornata internazionale in memoria delle vittime della *Shoah*; il 10 febbraio, Giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, e il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra Nazione nel mondo libero e democratico; poi anche il 9 novembre, cari colleghi, il Giorno della libertà, quale ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino. Il 25 aprile, la prima data che ho citato, deve diventare la festa della riconciliazione, come peraltro ci ha insegnato il presidente Ciampi, nominato poc'anzi dal senatore Verini, il quale, pur partigiano, disse nel 2001: «Abbiamo sempre presente, nel nostro operare quotidiano, l'importanza del valore dell'unità dell'Italia. Questa unità che sentiamo essenziale per noi, quell'unità che, in fondo oggi, a mezzo secolo di distanza» lo diceva nel 2001 «dobbiamo pur dirlo, era il sentimento che animò molti dei giovani che allora fecero scelte diverse: che le fecero credendo di servire ugualmente l'onore della propria Patria».

di uno stravolgimento rispetto al suo significato originale. La particolarità «consiste nel fatto che qui da noi l'antifascismo, invece di rappresentare un elemento unificante tra destra e sinistra ha costituito viceversa un tratto divisivo tra le due. Ma ciò è accaduto (...) non perché i "moderati" italiani, la destra, non siano abbastanza antifascisti. Ma soprattutto perché essi non vogliono esserlo al modo che vorrebbe la sinistra». «Non bisogna dimenticare che dietro di esse, quando si parla di queste cose, c'è una lunga storia, nel corso della quale, per l'appunto, un partito che si chiamava Partito comunista non solo usò a lungo la sua massiccia partecipazione alla Resistenza, la sua adesione all'antifascismo, per quasi identificarsi con esso e in tal modo cercare di far dimenticare le proprie scarse credenziali democratiche, ma per molto tempo ebbe pure l'abitudine di qualificare come "fascista" qualunque "moderato" che combattesse con decisione i suoi disegni, pretendendo che in nome dell'antifascismo ogni "onesto democratico" facesse altrettanto. *(Applausi)*. che quello che invece non si adeguasse rischiava facilmente che l'antifascismo fosse usato contro di lui». Vedete, queste parole che ho usato non sono le parole del senatore Speranzon o di un esponente della destra politica italiana, ma di Ernesto Galli della Loggia. L'antifascismo non può essere usato come arma retorica per screditare l'avversario politico o distribuire patenti di democraticità a questo o a quel partito nel Dopoguerra. Caro collega Verini, ci sono state moltissime occasioni in cui si è abusato del termine antifascismo, arrivando a compiere nel suo nome atti di efferata violenza come il rogo di Primavalle, che è stato commemorato qualche giorno fa da lei stesso in quest'Aula. agli innumerevoli omicidi delle Brigate rosse. Come non ricordare poi che quel Muro di Berlino di cui con la nostra mozione chiediamo il ricordo il 9 novembre si chiamava si chiamava *antifaschistische schutzwall*, muro di protezione antifascista, forse perché i comunisti, di là della Cortina di ferro, ritenevano che Willy Brandt e la socialdemocrazia della Repubblica federale

non hanno votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo che condanna ogni potere totalitario, compreso il comunismo. È comoda la chiave di lettura della della sinistra che, ogni qualvolta si tratta di parlare di comunismo, evita di usare quella parola e - come ha fatto adesso il senatore Verini - parla di stalinismo, maoismo e

risoluzione che condanna tutti i totalitarismi rappresenti qualcosa di indecente. *(Applausi)*. Noi lezioni di democrazia da chi non condanna ogni totalitarismo non le accettiamo. E forse è il caso che cominciate a leggere la Costituzione italiana,

Se voi non voterete la nostra mozione, è del tutto evidente che la Costituzione italiana non solo non l'avete letta, ma soprattutto non l'avete compresa. Dico al senatore Verini e al senatore Speranzon che non è colpa mia se il Regolamento prevede solo cinque minuti per illustrare

Lasciatemi ricordare Vladimir Kara-Murza, appena condannato a venticinque anni di prigione nelle carceri di Putin; Alexey Navalny, che sempre in quelle prigioni sta marcendo. È bello e giusto che il nostro Paese si schieri senza infingimenti e senza tentennamenti contro tutti i totalitarismi *(Applausi)* e celebri tutte le date che ci hanno condotto a essere una Nazione. Penso però che qualche volta provare a diluire una situazione dentro a tante altre situazioni simili faccia perdere di vista l'obiettivo. Voglio cioè dire Voglio cioè dire che, tra tutti i totalitarismi che purtroppo hanno macchiato la storia dell'umanità, ce n'è uno che sul nostro Paese ha lasciato i segni nella carne, nel sangue e nella storia. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Noi siamo figli di una storia particolare, nella quale il totalitarismo, con le sue mille facce, si è manifestato in questo Paese nella forma del fascismo. Non possiamo ignorarlo. Non possiamo pensare che per un italiano tutti i totalitarismi siano proprio uguali, perché c'è la differenza che c'è con una malattia. Siamo contro tutte le malattie e siamo solidali con chiunque abbia una malattia, ma, se una malattia ha ucciso un nostro congiunto, se proprio quella malattia ha toccato toccato la carne viva della nostra famiglia, noi forse ci iscriveremo all'associazione di quei malati e sosterremo la ricerca in particolare contro quella malattia. È normale. Quando infatti una cosa tocca la tua storia, ti tocca personalmente,

che il 17 marzo diventarono Re d'Italia, anziché Re di Sardegna e del Piemonte, sono gli stessi che, nel 1938, firmarono le leggi razziste e razziali che ancora oggi macchiano la storia della nostra Patria. È per questo che penso che dobbiamo fare uno sforzo importante, perché poi, da quella storia, è nata anche la nostra Repubblica. Se oggi siamo qui, cari colleghi, è in parte anche perché il 17 marzo è nato il Regno d'Italia. In quest'Aula sedevano i senatori del Regno,

perché il tacco nazista non si sollevasse e non levasse il giogo sotto il quale il nostro Paese era finito; e c'erano italiani grazie ai quali si è scritta la Costituzione e grazie ai quali anche culture politiche che quella Costituzione non hanno scritto oggi legittimamente governano questo Paese. *(Applausi)*. È per questo che penso che questa debba essere la festa di tutti, che debba essere la festa dell'antifascismo, perché il fascismo è il contrario della democrazia e noi siamo qui, cari colleghi, perché, grazie al cielo, in questo Paese ha vinto la democrazia. Io mi aspetto che celebriamo tutte le feste e quindi sono d'accordo sul 17 marzo come sulla data della caduta del Muro di Berlino: sono tutte date importanti, ma se ce n'è una che ha fatto di noi donne e uomini liberi, quella è il 25 aprile, la data nella quale le forze della democrazia hanno sconfitto quelle della tirannia, dell'oscurantismo, della violenza e dell'assenza di diritto. Viva la Repubblica italiana, antifascista, che ci dev'essere cara, carissima al cuore!

muoversi in maniera evidente contro ogni forma di totalitarismo ha un carattere che, in questa Aula, diventa fondamentale.

una storia collettiva, ma esistono anche storie individuali, cariche di sogni, di frustrazioni, di realtà scomode, anche nascoste, anche colpe. Non esiste persona pura non esiste persona che possa arrogarsi il diritto di rappresentare totalmente la verità e la purezza. Questa

che chi si crede giusto e puro totalmente è folle. *(Applausi)*. È folle, perché in ognuno di noi, certo in maniera diversa, spesso nascosta, esiste una realtà scomoda e imbarazzante, per la quale si tende a indicare la luna, la vecchia metafora, scordandosi il proprio naso e il proprio dito. Ecco perché mi stride chi

È assolutamente antistorica, antiumana e antievolutiva ogni forma di totalitarismo che non vuole salvare nulla. Il fascismo, ma anche il comunismo, è antievoluzione, è contro il nostro DNA, è contro quel mistero strano, affascinante e terribile che si chiama evoluzione, in cui spesso persino una disabilità, persino una malattia genetica, persino una contraddizione nella linearità del nostro percorso che si chiama storia, crea

della scienza che rappresento e per la quale non accetto lezioni da nessuno - siano persone dolcissime, piene d'amore, piene di attenzioni, che vivo anche nella mia famiglia allargata, e siano tentativi di evoluzione magari dal punto di vista dell'esempio, della tolleranza, dell'amore assoluto, della pazienza. Ebbene, con queste persone la maggior parte dei medici, che condanno - è la mia corporazione, è l'orgoglio della mia vita essere medico dopo il mio bisnonno - ha sbagliato. con mia madre, facendo partorire - io dico per fortuna, ma qualche volta mi arrabbio anche - una persona disabile, perché secondo lui la donna doveva partorire con dolore, perché così amava di più il figlio. Così mi ha fregato, perché sono nato asfittico forse è stato anche quello un tentativo di attenzione positiva; io ne avrei fatto volentieri a meno, ma questi sono affari miei.

che su temi come questi, il totalitarismo, quindi anche la diversità,

rotondi o quadrati, non ci può essere qualcuno che dà lezioni a qualcun altro. Vi giuro che sono pronto in qualsiasi momento a lasciare quest'Aula per sempre perché, nel momento in cui mi crederò incapace di assolvere al minimo compito per cui qualche cittadino mi ha delegato, non posso "fregare" le speranze, i dolci sogni, le attese della piccola gente,

che non stanno indietro, non ci stanno proprio *(Applausi)*, non hanno diritto di essere rappresentati perché non sanno che possono essere rappresentati. certamente ai milioni di persone con disabilità, anche mentale, fisica, povertà, sofferenze legate alla mancanza di lavoro, alla disoccupazione; ci vogliamo pensare? A questi non interessa minimamente da dove proveniamo e quali scelte facciamo; vogliono sapere se esistono o meno, perché tante volte ce ne scordiamo che dobbiamo rappresentare gli ultimi.

non possiamo accettare gruppi che legittimano gli altri insisto nel dire che nel totalitarismo, qualsiasi esso sia, io, noi, non accetto lezioni da nessuno, ma casomai discussioni. Mi permetto di dire infine che esiste un popolo di persone con disabilità che vive un olocausto quotidiano; migliaia di medici, nei quali mi rappresento e sono felice di vivere, dicono però che è meglio che non viva perché è diverso, è meglio che non nasca o che partecipi alla meraviglia della vita

la gran parte degli italiani di oggi non ha provato cosa significa la privazione della libertà. Solo i più anziani hanno un ricordo diretto del totalitarismo, dell'occupazione straniera, della guerra per la liberazione della nostra Patria. Siamo cresciuti con i ricordi di una generazione di italiani che non esitò a scegliere la libertà, anche a rischio della propria sicurezza, anche a rischio della propria vita. Il nostro Paese ha un debito inestinguibile verso quei tanti giovani che sacrificarono la vita negli anni più belli, per riscattare l'onore della Patria, per fedeltà a un giuramento, ma soprattutto per quel grande, splendido e indispensabile valore che è la libertà. Lo stesso debito di gratitudine lo abbiamo verso tutti quegli altri ragazzi che versarono il loro sangue nella campagna d'Italia. Senza di loro, il sacrificio dei nostri partigiani avrebbe rischiato di essere vano. Con rispetto dobbiamo ricordare oggi tutti i caduti, anche quelli che hanno combattuto dalla parte sbagliata, sacrificando in buona fede la propria vita ai propri ideali e a una causa già perduta. Questo non significa naturalmente neutralità o indifferenza. Noi siamo - tutti gli italiani liberi lo sono - dalla parte di chi ha combattuto per la nostra libertà, per la nostra dignità e per l'onore della nostra Patria. In questi anni la storia della Resistenza è stata approfondita e discussa. È un bene che sia successo. La Resistenza è, con il Risorgimento, uno dei valori fondanti della nostra Nazione, un ritorno alla tradizione di libertà. E la libertà è un diritto che viene prima delle leggi e dello Stato, perché è un diritto naturale che ci appartiene in quanto esseri umani. Una nazione libera, tuttavia, non ha bisogno di miti; come per il Risorgimento, occorre ricordare anche le pagine oscure della guerra civile, anche quelle nelle quali chi combatteva dalla parte giusta ha commesso degli errori e si è assunto delle colpe. È un esercizio di verità, è un esercizio di onestà, un esercizio che rende ancora più gloriosa la storia di coloro che invece hanno combattuto dalla parte giusta, con abnegazione e con tanto coraggio. In quel momento tanti italiani di fedi diverse, di diverse culture e di diverse estrazioni si unirono per seguire lo stesso grande sogno, quello della libertà. Vi erano fra loro persone e gruppi molto diversi. Vi era chi pensava soltanto alla libertà, chi sognava di instaurare un ordine sociale e politico diverso, chi si considerava legato a un giuramento di fedeltà alla monarchia. Ma tutti seppero accantonare le differenze, anche le più profonde, per combattere tutti insieme. I comunisti e i cattolici, i socialisti e i liberali, gli azionisti e i monarchici, di fronte a un dramma comune scrissero, ciascuno per la loro parte, una grande pagina della nostra storia, una pagina sulla quale si fonda la nostra Costituzione, sulla quale si fonda la nostra libertà. Benché frutto evidente di compromessi, la Costituzione repubblicana riuscì a conseguire due obiettivi nobili e fondamentali: garantire la libertà e creare le condizioni per uno sviluppo democratico del Paese. Non fu poco, anzi fu il miglior compromesso allora possibile. Oggi il nostro compito, il compito di tutti è quello di costruire finalmente un sentimento nazionale unito. Dobbiamo farlo tutti insieme, quale che sia l'appartenenza politica; tutti insieme per un nuovo inizio della nostra democrazia repubblicana, dove tutte le parti politiche si riconoscono nel valore più grande, che è appunto la libertà, e nel suo nome si confrontino per il bene e nell'interesse di tutti. L'anniversario della riconquista della libertà è dunque l'occasione per riflettere sul passato, ma anche per riflettere sul presente e sull'avvenire dell'Italia. Se riusciremo a farlo insieme, avremo reso davvero un grande servizio non a una parte politica o all'altra, ma al popolo italiano e soprattutto ai nostri figli, che hanno il diritto di vivere in una democrazia finalmente pacificata. Noi abbiamo sempre respinto la tesi che il nostro avversario fosse il nostro nemico: ce lo imponeva e ce lo impone la nostra religione della libertà. Con lo stesso spirito siamo convinti che siano maturi i tempi perché la festa della Liberazione possa diventare la festa della libertà e possa togliere a questa ricorrenza il carattere di contrapposizione che la cultura rivoluzionaria le ha dato e che ancora divide piuttosto che unire. Il 25 aprile fu all'origine di una nuova stagione di democrazia e in democrazia il voto del popolo merita l'assoluto rispetto da parte di tutti. Il popolo, dopo il 25 aprile, votò pacificamente per la Repubblica e la monarchia accettò il giudizio popolare. Poco dopo, il 18 aprile 1948, la scelta popolare fu di nuovo decisiva per il nostro Paese:

L'Italia divenne parte dell'Europa e dell'Occidente, fu tra i promotori dell'unità atlantica e dell'unità europea; un Paese reietto divenne un Paese rispettato. Oggi i nostri giovani hanno davanti a loro altre sfide: difendere la libertà conquistata dai loro padri e ampliarla sempre di più, consapevoli, come sono, che senza libertà non vi può essere né pace, né giustizia, né benessere. È proprio nei confronti degli eroi di allora e di oggi che noi tutti abbiamo una grande responsabilità: quella di mettere da parte ogni polemica, di guardare all'interesse della Nazione, di tutelare il grande patrimonio di libertà che abbiamo ereditato dai nostri padri. abbiamo la responsabilità e il dovere di costruire per tutti un futuro di prosperità, di sicurezza, di pace e di libertà. Viva il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi! Come avranno compreso i più attenti, mi sono limitata a citare ampi stralci dell'intervento del presidente Silvio Berlusconi nel 2009 a Onna. A lui, che in questi giorni è in ospedale, va il nostro saluto più cordiale, il ringraziamento per la sua sapienza e lungimiranza e il miglior augurio in occasione del prossimo 25 aprile, che è la festa di tutti gli italiani.

Presidente, l'Aula del Senato della Repubblica, così come quella della Camera dei deputati, è luogo simbolo della nostra democrazia: qui noi agiamo da uomini liberi, forti ognuno delle proprie convinzioni, della possibilità di battersi per esse senza costrizioni. Questa libertà e questa eguaglianza sono scritte nella nostra Costituzione

abbiamo il dovere di onorare ogni giorno parlamentari martiri dell'antifascismo, come Giacomo Matteotti, come Giuseppe Di Vagno, come Antonio Gramsci. Ogni volta che entro in quest'Aula sento la responsabilità verso le donne e gli uomini della Resistenza che seppero riconquistare per tutti noi la libertà e la democrazia che il fascismo aveva infamato e ucciso. Ci sono parole che sono sacre per la nostra Repubblica, come quelle di Piero Calamandrei rivolte ai giovani: «se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati». *(Applausi)*. La Resistenza e l'antifascismo sono il fondamento della nostra Repubblica e il 25 aprile è la festa più bella e la più importante e non è la festa di alcuni. Com'è stato detto anche in quest'Aula, è la festa che unisce tutti gli italiani, come ha unito e deve unire tutti gli italiani, perché è la Festa della liberazione dal nazifascismo, dalla dittatura, dall'occupazione. È la festa più patriottica: quelli che noi chiamiamo e abbiamo chiamato partigiani, tra loro, durante la lotta di liberazione, si chiamavano patrioti. E fu lotta patriottica per riscattare dal fascismo il nome nostro, dell'Italia. la Resistenza fu armata e fu civile: contadini o cittadini che nascosero nelle loro case un antifascista o un ebreo, mettendo a rischio non solo la propria vita, ma quella dell'intera famiglia, e il più delle delle volte non per comunanza politica o convinzione ideologica, ma per il sentimento innato di umanità e di fratellanza, per la volontà di non rassegnarsi all'ingiustizia, alla ferocia, al destino e alla sopraffazione. Ecco perché la Resistenza appartiene a tutti e noi abbiamo il dovere di coltivare una memoria condivisa e di trasmetterla alle nuove generazioni, per cementare lo spirito repubblicano e per farlo non dobbiamo mai, per alcun motivo, mistificare la parte del torto e quella della ragione *(Applausi)*, fare finta di non sapere l'abisso che divide libertà e dittatura. La sintesi più efficace di tutto questo venne data, appunto, anni fa in un dibattito pubblico da Vittorio Foa, che fu partigiano, nei confronti di un parlamentare missino che era stato volontario a Salò con Mussolini, al quale Foa disse: «Se avesse vinto lei, io sarei ancora in prigione. Avendo vinto io, lei è senatore della Repubblica e può parlare qui con me». I valori e gli ideali della Resistenza sono le basi storiche e morali della nostra Repubblica e il legame di legittimazione che unisce in un patto civico memoria e futuro, come abbiamo scritto nella nostra mozione. però - lo vediamo - c'è un tentativo smaccato e inaccettabile di erodere questo patto e da qui la nostra mozione. mozione. Presidente Gasparri, per suo tramite mi voglio rivolgere al presidente La Russa, che mi dispiace non sia qui in questo momento. Signor presidente La Russa, sono insopportabili la continua provocazione, la mistificazione, lo scherno sulla memoria della Resistenza, che è sacra a quest'Assemblea e a tutti gli italiani, perché riguarda il sacrificio e il testamento di 100.000 e 100.000 morti ed è cuore pulsante, non un dibattito accademico o teorico. Presidente La Russa, tutti sanno ciò che avvenne a via Rasella *(Applausi)*, in uno degli atti più importanti della Resistenza militare italiana, un atto di guerra legittimo contro l'invasore. Tutti sanno ciò che avvenne, presidente La Russa, e lo sa anche lei; eppure deliberatamente ha voluto far credere che ad essere colpita fosse - e cito le sue parole - «una banda musicale di semipensionati». Presidente La Russa, se un ragazzo, ascoltando questa versione data dalla seconda carica dello Stato, pensasse che i cattivi siano stati i partigiani a prendersela con dei musicisti, come potremmo biasimarlo? signor Presidente, stanno qui la falsificazione, il negazionismo subdolo, l'oltraggio che noi non possiamo accettare. Non può esserci mai mistificazione, mai! Non può esserci sulla Resistenza, non può esserci da parte di chi ha incarichi istituzionali, non può esserci da parte della seconda carica dello Stato. E la risposta più netta lei, presidente La Russa, l'ha avuta da Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica romana, che ha detto, sono sue parole: «Non erano musicisti, erano soldati delle SS naziste che occupavano il Paese con la complicità dei fascisti e che deportavano gli ebrei nei campi di sterminio». Ha continuato Ruth Dureghello: «Viva i partigiani, che hanno messo a rischio la propria vita per restituire libertà e sovranità, all'Italia». Queste le sue parole. Via Rasella fu un atto di guerra legittimo. Sui muri, all'incrocio tra via Rasella e via del Boccaccio, ci sono ancora i fori dell'attentato, che non sono mai stati cancellati per volere della popolazione di quel di quel quartiere, perché quei fori sono impronte della storia. Lei sa, signor Presidente, che Carla Capponi e Rosario Bentivegna, partigiani a via Rasella, sono stati insigniti delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare. L'indomani, alle Fosse ardeatine, 335 innocenti furono vittime dell'ignobile rappresaglia nazista. Non furono uccisi,

che quei 335 martiri non furono uccisi perché italiani, ma perché antifascisti o ebrei, uccisi da altri italiani, perché una delle liste delle persone massacrate alle Fosse ardeatine fu consegnata ai tedeschi dai fascisti italiani. È la storia,

voleva la dittatura. C'è in questo un tentativo di denigrare l'intera Resistenza, operando un rovesciamento della verità storica e cioè che i comunisti italiani, al pari delle altre forze antifasciste, furono i fondatori della nostra Repubblica, i costruttori e i difensori - sempre, in ogni circostanza, anche la più terribile ed eversiva della nostra democrazia e qui lo dobbiamo affermare. Per questo tutti noi dobbiamo la conquista della libertà, che la tirannide fascista aveva ucciso, e la Costituzione italiana a queste forze. Quella Costituzione firmata dal presidente De Gasperi, dal presidente Einaudi e, insieme a loro, da Umberto Terracini, un comunista italiano, presidente dell'Assemblea costituente. Chiediamo rispetto per la storia del nostro Paese: a questo sacrificio che oggi ognuno di noi e la seconda carica dello Stato possono sedere ai vertici della nostra Repubblica. Signor Presidente, mi avvio Siamo parte di una storia che è più grande di noi e il 25 aprile ne è l'emblema, data fondativa della Repubblica; la Resistenza, come il Risorgimento lo ha detto il presidente Mattarella - con gli stessi «ideali di libertà, umanità, civiltà e fratellanza». Non c'è futuro senza il dovere della memoria e senza il dovere della verità storica, che, solo se rispettata, è maestra per tutti. La tensione civile e morale dei valori dell'antifascismo è l'essenza stessa della democrazia, in Italia e in ogni parte del mondo, ed è nostro dovere trasmetterla alle nuove generazioni. *(Applausi)*.

discutiamo di memoria, ricorrenze e commemorazioni storiche. Per affrontare questi temi è essenziale una certa onestà intellettuale. Fra pochi giorni celebreremo la ricorrenza del 25 aprile. È impensabile non tracciare un legame tra la liberazione dal nazifascismo e ciò che furono i suoi frutti: la Costituzione e la Repubblica. Come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Carta costituzionale è il fondamento saldo e vigoroso della nostra unità nazionale. I suoi principi e i suoi valori sono nel DNA della nostra democrazia. Lancio oggi un appello dai banchi di quest'Aula. Gli italiani che ci guardano là fuori non meritano che la politica si divida. Ogni anno c'è un pretesto per trasformare questa ricorrenza in una festa della divisione. È successo persino durante l'emergenza Covid e con un Governo di unità nazionale. Quest'anno cosa accadrà? Agitare la bandiera della strumentalizzazione nel tentativo di indebolire la maggioranza e questo Governo non solo è un errore, ma rischia seriamente di impoverire il dibattito politico e culturale di questo Paese. Un attimo dopo, senza uno sforzo di condivisione, avremmo due opposte tifoserie. Sarebbe deleterio. Sarebbe sbagliato portare sul campo della contrapposizione politica temi fondanti della nostra democrazia. *(Applausi)*. Sarebbe pericoloso, visto che parliamo di memoria storica e di valori come la libertà. Su questi temi noi della maggioranza lanciamo un messaggio di pacificazione da questi banchi. Il nostro invito è di astenersi da qualsiasi tentativo di delegittimazione preventiva. Dal *premier* Meloni, in occasione dell'insediamento del Governo e della fiducia alle Camere, arrivarono parole inequivocabili: «Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi non democratici, per nessun regime, fascismo compreso. Ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna». Il 25 aprile non è un feudo identitario della destra o della sinistra. Non ha senso dire che è una festa di tutti e poi un minuto dopo delegittimare l'avversario. La nostra storia ha avuto un punto di frattura certamente nell'antifascismo, che per noi è l'elemento fondante della nostra Repubblica, quindi contro tutte le dittature e i totalitarismi. *(Applausi)*. Nessuno, men che meno la sinistra, può arrogarsi il diritto di appropriarsi della cultura antifascista, cultura e valori antifascisti che sono presenti dalla prima all'ultima pagina della nostra bellissima Costituzione. La memoria, onestamente coltivata, altrettanto onestamente ci fa agire nel presente. Questo vuol dire pacificazione. Cari colleghi, il 25 aprile non è la casa di una o dell'altra parte politica, ma è la casa di tutti, così come lo sono le altre ricorrenze storiche che ricordano i momenti fondamentali della storia dell'Italia, unita, libera e democratica; il 1° maggio, Festa del lavoro; il 2 giugno, nascita della Repubblica ed elezione dell'Assemblea costituente; il 17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia; il 4 novembre, Festa dell'unità delle Forze e altre date significative della nostra storia, come ad esempio il 27 gennaio, Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah *(Applausi)*; il 10 febbraio, il massacro delle Foibe; il 18 aprile; il 9 novembre, giorno in cui cadde il Muro di Berlino, che pose fine alla guerra fredda. La pacificazione è una strada possibile? Per noi sì, non può non essere che così. Rispettare i valori costituzionali di unità e di libertà seguendo lo spirito repubblicano e accogliendo i richiami più volte manifestati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, sull'importanza del ricordo a prescindere da qualsiasi ideologia. Sono questi per noi della maggioranza di centrodestra i principi che ci ispirano e che oggi in quest'Aula ci spingono a lanciare un appello a tutte le forze politiche: deponiamo le armi ideologiche, solo così apriremo la strada alla pacificazione nazionale. Per queste ragioni,

in quest'Aula dalla senatrice Segre, il primo giorno della legislatura, come una vera e propria pietra miliare, ma temo che non siano state sufficientemente comprese e assimilate come meritano. Quelle parole non ripetono - come pure spesso è necessario fare - cose che sono state già dette, ma indicano, invece, una strada per superare, pur nel quadro della contrapposizione democratica tra visioni e progetti alternativi, lacerazioni che non sono mai state superate del tutto e che continuano spesso a inquinare la dialettica democratica di questo Paese. Vi sono date che non sono semplicemente ricorrenze, ma che devono essere vissute come riti fondativi di una Repubblica basata su valori che tutti condividono. La senatrice Segre ne indicò tre: la Festa della liberazione, quella del lavoro e quella della Repubblica. Non sono ricorrenze qualsiasi e sono diverse da ogni altra data. Sono i pilastri su cui si basa la Repubblica democratica fondata sul lavoro. Dunque, sono valori che possono e devono accomunare, non dividere e contrapporre, ma perché questo possa realizzarsi è necessario che ci siano limpida chiarezza e massimo rispetto per la verità storica. Quelle date sono così importanti proprio perché racchiudono e sintetizzano l'eredità di una esperienza storica che non può essere contraffatta, non può essere edulcorata, non può essere raccontata da ciascuno a modo suo. Il dovere delle istituzioni è seguire la rotta indicata quel giorno dalla senatrice Segre e farlo garantendo quel rispetto essenziale per la verità storica.

Voglio dirlo con la massima calma, senza toni da comizio e, tuttavia, con tutta la chiarezza possibile. Le parole pronunciate dal Presidente del Senato in occasione dell'anniversario del massacro nazista delle Fosse ardeatine hanno offeso la verità storica e hanno offeso gli italiani, tutti gli italiani, non solo quelli che hanno votato per la mia parte politica. *(Applausi)*. È stato un insulto ai danni della verità storica far passare un atto di guerra contro l'invasore per un agguato vigliacco ai danni di una banda di pensionati. I soldati del reggimento di polizia Bozen uccisi dai patrioti in via Rasella non erano pensionati e non erano una banda musicale. Erano parte di un esercito invasore, che per nove mesi, dal 10 settembre del 1943 al 4 giugno 1944, strinse Roma in una morsa di terrore. Io so che il Presidente del Senato di quelle frasi si è scusato, ma ci sono volte che, per scusarsi, non bastano le parole e servono, invece, i gesti; gesti che, evidentemente, non ci sono stati. In quei mesi, a Roma, tutti erano terrorizzati. Erano terrorizzati gli ebrei che, dopo la razzia del 16 ottobre nel Ghetto, che contò 1.023 deportati portati a morire nei campi di sterminio, potevano essere riconosciuti e mandati a morire ogni giorno. Erano terrorizzati i cittadini, che potevano essere deportati in massa in Germania a fare da schiavi, come avvenne nel rastrellamento del Quadraro il 17 aprile del 1944. Erano terrorizzati i Carabinieri: 1.500 di loro furono deportati. Erano terrorizzati gli antifascisti, torturati dai tedeschi e dai collaborazionisti francesi in via Tasso, dove furono martoriate oltre duemila persone, ma anche a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Jaccarino, dalla banda Koch, e nei sotterranei di Palazzo Braschi dalla banda Bardi. Erano terrorizzate le donne, falciate mentre protestavano per la penuria del pane al ponte dell'Industria, il 7 Aprile 1944. E a seminare terrore erano non solo gli occupanti tedeschi, ma anche i fascisti collaborazionisti italiani, come ha ricordato da Auschwitz il presidente Mattarella. Questa era la Roma delle Fosse ardeatine. Questa era la Roma occupata dal brutale esercito di Hitler e dai collaborazionisti schierati con l'invasore. Roma in quel momento però è anche la città nella quale c'è una fortissima resistenza; una città in cui la vita non ha nulla di normale; una città in cui si combatte, in cui anche Centocelle è stata appena rastrellata, in cui ci sono le fucilazioni come a Forte Bravetta. di azione patriottica (GAP) che presero le armi lo fecero come fa sempre, ovunque, chi è costretto a combattere in una città occupata. Questa è la verità storica e non la si può addomesticare. *(Applausi)*. Credo che quella versione bugiarda della storia sia stata davvero un'offesa per tutti gli italiani. Cosa spinse i combattenti dei GAP e delle formazioni partigiane a rischiare la vita e la tortura? I nazisti avrebbero perso la guerra: ormai cominciava ad essere chiaro a tutti in quei mesi. Gli alleati erano alle porte di Roma ed era inevitabile che cacciassero presto gli occupanti tedeschi. E allora perché tante donne e tanti uomini non se ne rimasero semplicemente nascosti ad aspettare la liberazione? Per velocizzare la liberazione, certamente, ma anche perché non volevano che la libertà dell'Italia fosse solo un regalo degli eserciti alleati. La posta in gioco non era soltanto qualche settimana di occupazione in più, ma erano la dignità e l'onore dell'Italia, il suo riscatto, la sua possibilità di diventare padrona del proprio destino democratico. E, anche se ci fu chi combatté dalla parte sbagliata per un malinteso, ma sincero, senso dell'onore, questo non cambia il senso delle cose e della storia. Furono solo i partigiani a riscattare l'onore e la dignità di tutto il Paese. Ed è solo con questa solida consapevolezza alle spalle che possiamo incamminarci sul percorso che ci ha indicato la senatrice Segre.

noi del Gruppo per le Autonomie - come sapete - siamo particolarmente legati al concetto di rappresentanza del territorio da cui proveniamo e quindi abbiamo il dovere di tener conto dei sentimenti anche un po' particolari che hanno le minoranze linguistiche che abitano nei territori con le autonomie speciali che la nostra Repubblica ha ritenuto di riconoscere. Ho personalmente molto apprezzato la sincerità con cui il senatore Speranzon ha espresso le convinzioni della sua parte politica a sostegno della mozione che ha presentato. Credo che questa sincerità sia il punto di partenza per superare le cesure, le incomprensioni e le differenze di vedute tuttora presenti, anche a volte artificiosamente accentuate per scelta politica, riguardo alle feste che rappresentano o che dovrebbero rappresentare l'unità del nostro Paese. La nostra Costituzione - è già stato detto - affonda le sue radici nella negazione del fascismo, perché è stata redatta in un momento in cui era appena finita la dittatura fascista e quindi doveva prenderne le distanze. Lo ha fatto in diversi passaggi, come all'articolo 3, che ricorda l'abominio delle leggi razziali; all'articolo 6, che ricorda le persecuzioni contro le minoranze tedesche, latine, francesi e slovene; mentre l'articolo 10 fa riferimento indirettamente all'isolamento dell'Italia uscita dalla Società delle Nazioni; l'articolo 11 ricorda la tragedia della Seconda guerra mondiale e delle infauste guerre

tantissimi riferimenti, nella nostra Costituzione, a quello che accadde nel ventennio e che non deve più verificarsi. Devo dire che la comunità da cui provengo ha vissuto in maniera particolarmente forte la sofferenza di sottostare a un regime a un regime fascista che ha impedito alla minoranza tedesca dell'Alto Adige di usare pubblicamente la sua lingua e che ha costretto questa minoranza a inventarsi forme illegali per continuare a portare avanti la propria identità culturale e la propria lingua.

purtroppo, per quanto mi riguarda - non potrà avere il mio voto favorevole, perché non c'è la parola antifascista e io non posso permettermi di rappresentare il mio territorio senza che ci sia quella parola. Lo devo dire molto chiaramente. Il Gruppo Per le Autonomie ha invece sostenuto fortemente la mozione presentata dalla nostra parte politica, perché siamo convinti che i valori comuni che abbiamo si riconducono al valore dell'antifascismo che presiede la Festa del 25 aprile. Ricordo una citazione di Gianfranco Fini, uno dei padri della destra moderna italiana, secondo cui non c'è stata una destra in grado di dire che ci riconosciamo in pieno nei valori antifascisti, ma la destra politica italiana e, a maggior ragione, i giovani devono senza ambiguità dire alto e forte che si riconoscono in alcuni valori presenti nella nostra Costituzione, come libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale. Sono valori che hanno guidato il cammino politico della destra e quindi bisogna ribadire che la destra vi si riconosce: è un atto doveroso. Lo disse Gianfranco Fini. Quello che disse Berlusconi a Onna è già stato ricordato, quindi non lo ripeterò, ma è evidente che c'è stata - anche in esponenti di spicco della destra italiana - una presa di posizione chiarissima contro il fascismo, che non toglie che si debba essere contro tutti i totalitarismi. Signori, è assolutamente chiaro: il mondo va sempre più in una direzione in cui siamo divisi tra Paesi dove ci sono Governi democraticamente eletti e Paesi dove ci sono Governi assolutisti, che sono stati nominati attraverso percorsi non di democrazia. Non possiamo che stare dalla nostra parte e, quindi, quindi, assolutamente riconosco il diritto di chi governa oggi l'Italia di portare avanti le sue idee, perché credo profondamente nella democrazia che fa sì che chi la pensa diversamente da me, se ha la maggioranza, possa portare avanti le sue idee. Questo lo devo dire in modo molto chiaro contro i totalitarismi, come detto, ma non posso neanche accettare che vengano fatte mistificazioni della storia. Qualcuno sostiene che la Resistenza non era dovuta; anzi, è stato un episodio di secondo piano del del Dopoguerra o della fase finale della Seconda guerra mondiale. Signori, però i partigiani hanno combattuto una loro guerra contro l'oppressore che rientra nel pieno diritto di ogni popolazione di difendersi quando viene invasa, come succede adesso Un'altra mistificazione che ogni tanto salta fuori è che la Resistenza non aveva importanza militare e quindi è stato in fondo un episodio irrilevante, ma non è vero, perché la Resistenza italiana è stata una spina nel fianco per gli occupanti tedeschi e per la Repubblica di Salò. I dati che si evincono dai rapporti di gerarchi repubblichini e dalle memorie dei generali tedeschi affermano questo e dicono che nel Nord Italia i nazifascisti impiegarono parecchie divisioni, sebbene di seconda categoria, che però vennero distolte da altri fronti per combattere i nostri partigiani e anche a Roma i tedeschi incontrarono difficoltà. Il maresciallo Kesselring, durante il suo processo, affermò che Roma fu, tra tutti i Paesi occupati, la capitale che più diede problemi e dove era impossibile mandare le truppe in licenza dal fronte per riprendersi e riposarsi. Il generale Alexander, comandante di tutte le truppe alleate del Mediterraneo, disse che aveva cominciato a rispettare gli italiani dopo che aveva scoperto come i partigiani avevano sfidato a Roma un battaglione tedesco armato. armato. Prendiamo anche atto che la Resistenza ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione dell'Italia di oggi e di quello che noi oggi siamo, sulla base della Costituzione repubblicana. Presidente, l'Italia è una, ma è una democrazia per cui è legittimo avere opinioni divergenti; se c'è però una parte, sia pure nostalgica e minoritaria, che punta a spezzare il legame tra antifascismo e istituzioni, che mette sullo stesso piano gli afflati di libertà e uguaglianza con le ideologie totalitarie che hanno portato dolore e distruzione, va respinta con la massima forza. Soprattutto non può trovare riparo, neppure sotto forma di sgrammaticatura istituzionale, nel cuore delle nostre istituzioni, che invece devono sempre essere protese a ribadire il più sacro dei concetti. è una festa di tutti ed è la festa fondamentale sulla base della quale è nata la Repubblica italiana, in cui viviamo oggi. Dobbiamo esserle grati e dobbiamo essere grati a tutti quelli che hanno contribuito, a quel tempo, a farci diventare quello che siamo.

che ci conducono al cuore stesso dell'articolo 1 della nostra Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Devono essere vissute pertanto con autentico spirito repubblicano; non possono e non devono essere divisive. Noi oggi ci presentiamo qui con due mozioni diverse. Questa è una prima sconfitta e lo dico con amarezza. Penso che, di fronte a una mozione presentata dalla minoranza, il cui centro principale era il tema del 25 aprile, probabilmente si sarebbe potuto fare lo sforzo della costruzione comune di un testo. È l'idea stessa che magari si possa votare quel testo, ma che non ci si possa riconoscere con un atto comune di questo Parlamento, a determinare una sconfitta in sé, della quale ognuno di noi porta un pezzo di responsabilità, ma che oggi in qualche modo voglio richiamare all'attenzione di tutti voi. La piena condivisione delle feste nazionali di questo nostro calendario civile scandisce un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, e può, anzi deve aprire a gesti nuovi e inattesi. Sul tappeto c'è non una sterile divisione sul passato, ma la necessità di un continuo rinnovamento di quel patto democratico e repubblicano che può e deve dare forza alla nostra democrazia e alle nuove sfide che abbiamo di fronte.

più forte, più capace di trarre forza proprio dal fare una volta per tutte i conti con la storia di questo Paese e inverare una fattiva condivisione dei valori che stanno alla base della convivenza civile: i valori dell'antifascismo. È un dovere - fatemelo dire anche in questo caso - innanzitutto di chi ha la responsabilità di Governo, di smettere una volta per tutte ambiguità sterili, atteggiamenti animati da incomprensibili definizioni legate a qualche revanscismo. Ha fatto bene la collega a citare una pagina che io reputo importante della nostra vita democratica, cioè il 2009 a Onna. Il presidente Berlusconi in quella circostanza tentò un autentico gesto di pacificazione *(Applausi)*, che io voglio riconoscere oggi e legare a un saluto e a un apprezzamento di quello che ha fatto e di quello che probabilmente quest'Assemblea ancora deve interpretare. È per questa ragione che che io non ho capito come mai dentro la vostra mozione non c'è mai, neppure una volta, la parola "antifascismo".

presentata dalla minoranza, ma non posso negarvi che a quel gesto di pacificazione a Onna di Berlusconi oggi probabilmente avrebbe dovuto corrispondere una parola netta scritta anche sulla mozione *(Applausi)* nella quale voi avete identificato una serie di date, tutte importanti, tutte fondamentali, ma che a mio modo di vedere dovevano portare o alla costruzione di un testo condiviso oppure a una nettezza nell'indicazione di quella parola ("antifascismo") a cui vi richiamavo. richiamavo. La nostra Repubblica è nata dalla lotta di liberazione del Paese dall'oppressione nazifascista. Il 25 aprile è una data fondativa della nostra democrazia, di ricomposizione dell'unità nazionale; la straordinaria conquista della libertà, dell'affermazione del proprio diritto alla pace, dopo la guerra voluta dal regime fascista, dopo il prezzo altissimo pagato dalle popolazioni civili con la brutalità delle rappresaglie, dopo l'indicibile violenza contro l'umanità, con crimini terribili culminati nella Shoah. Non può essere nascosta, non può essere lasciata alla nostra mozione: dev'essere scritta da parte di tutti. Questo è il punto. Ritengo pertanto che noi oggi noi oggi avevamo un'opportunità importante, perché siamo immersi in uno di quei periodi che vengono definiti tornanti della storia. Le nostre democrazie sono sotto attacco da parte delle autocrazie (Russia, Iran, Cina), che rifiutano quei valori che sono alla base della convivenza civile delle nostre società, che vogliono destabilizzarli e cancellarli. *(Applausi)*. È per questo che la risposta che noi diamo in termini di verità storica rispetto a quello che è accaduto al nostro Paese - come diceva molto bene il collega Scalfarotto - è oggi più che mai importante. Bernardo di Chartres che noi siamo come nani sulle spalle di giganti, cosicché possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'acume di vista o per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. Quei giganti possono consentirci di costruire un futuro di nuova forza per la nostra democrazia, senza polemiche inutili e sterili. e sterili. Quelli che noi dobbiamo guardare con gli occhi dei giganti sono i valori di libertà, giustizia, uguaglianza, rispetto dei diritti dell'uomo. E quelle tre date indicate all'interno della nostra mozione li simboleggiano a pieno. *(Applausi)*. per una memoria viva e operante è una battaglia di giustizia e di civiltà per nulla scontata, che passa per il riconoscimento e la celebrazione di quelle tre date fondative, di quelle tre feste civili che racchiudono il *pantheon* valoriale a cui noi dobbiamo necessariamente fare riferimento.

non c'è nulla all'interno di quelle date che non possa essere condiviso, ma mancano due punti fondamentali. Il primo è l'accettazione di un percorso comune

su un livello di assenza quasi totale di polemica, perché lo penserei sbagliato e inutile per la fase che sta vivendo il Paese *(Applausi),* con una bellissima citazione di Etty Hillesum che penso meriti di essere citata in quest'Aula: trovo bella la vita e mi sento libera. I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. La vita è difficile, ma non è grave. Dobbiamo prendere sul serio il nostro lato serio e il resto verrà allora da sé. Lavorare su sé stessi non è proprio una forma di individualismo malaticcio. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà trovata da ognuno di noi in se stesso, se ogni uomo sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e lo avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga, in amore, se non è chiedere troppo. Io non ho la pretesa che la discussione tra di noi possa trasformarsi in amore, ma ho la pretesa che in un'Aula parlamentare, dopo così tanti anni, si condividano insieme valori e principi importanti ed è la sfida che abbiamo di fronte nei prossimi anni.

siano state accompagnate da qualche polemica di troppo, forse perché per la prima volta nella storia un esponente della destra ricopre la carica di Presidente del Consiglio. L'auspicio di entrambe le mozioni oggi all'esame del Senato, di cui condivido la lettera e lo spirito e su cui il Gruppo Forza Italia voterà favorevolmente, è che le tensioni una volta per tutte si stemperino e si possano vivere tutte le ricorrenze nazionali con spirito patriottico e unitario, come tante volte auspicato anche dal presidente Mattarella. Non è purtroppo sempre così. Il nostro Paese vive un'anomalia rispetto alle principali democrazie occidentali. Non c'è ancora una memoria storica condivisa sugli eventi del Novecento, che in troppe occasioni vengono ancora trattati con spirito di parte - se mi consente, Presidente, un po' estremista - in una semplicistica contrapposizione fascismo-antifascismo. Alcune questioni sono restate tabù per troppo tempo e in questo senso ho molto apprezzato il dibattito che ha avuto luogo qualche giorno fa in quest'Aula sul rogo di Primavalle e la tragica morte dei fratelli Mattei.

senatori Verini, Mennuni e Gasparri. È questo lo spirito giusto con cui affrontare tematiche così delicate e trasmettere alle nuove generazioni, che quegli anni non hanno vissuto, una memoria condivisa di riconciliazione. Purtroppo, signor Presidente, le nuove generazioni non leggono Benedetto Croce, Piero Gobetti o Renzo De Felice. Temo che neppure guardino su RaiPlay trasmissioni come «La notte della Repubblica» o «Blu notte», che nel tempo hanno trattato i temi degli anni di piombo e del terrorismo. A quei giovani, che si informano solo sui *social*, una classe politica, responsabile e attenta, deve cercare di trasmettere valori autentici, democratici e di reciproco rispetto e giornate come quella in esame certamente potrebbero aiutare. Cercherò di affrontare i diversi temi posti oggi all'attenzione dell'Assemblea. Parto con un riferimento agli interventi del senatore Spagnolli e della senatrice Paita

oggi all'esame di quest'Assemblea, richiamando la risoluzione del Parlamento europeo del 2019, condanna senza riserve ogni regime autoritario, fascismo - e lo cita - nazismo, comunismo. non capisco quale sia la differenza semantica tra condanna del fascismo e antifascismo: francamente mi sfugge e credo di non sbagliare. Per questo innanzitutto oggi non possiamo non dirci antifascisti, se per antifascismo intendiamo condanna di quel regime illegale che cancellò le libertà democratiche del nostro Paese, si affermò con la violenza politica, si macchiò dell'infamia delle leggi razziali e trascinò l'Italia in una guerra disastrosa a fianco della Germania nazista. La resistenza al nazifascismo ci ha consegnato una Costituzione liberale, che rimane il nostro faro e la nostra bussola politica; un'Italia democratica e occidentale di cui dobbiamo essere orgogliosi, in cui siamo vissuti, abbiamo potuto studiare e affermarci professionalmente, coltivando i nostri ideali politici. Questo patrimonio di valori va difeso con le unghie e con i denti, tanto più in un drammatico momento storico in cui regimi autoritari, in cui chi critica lo Stato e la sua politica viene ucciso o messo in galera, sfidano in modo aspro i sistemi democratici. pari però, per un principio di riconciliazione nazionale e di memoria storica condivisa, non possono essere dimenticati altri episodi e le vittime innocenti di tanta insensata violenza politica, che purtroppo, anche nel dopoguerra, ha insanguinato il nostro Paese, senza per questo essere accusati di revisionismo o, peggio, di fascismo. Penso agli eccidi delle Foibe, al triangolo rosso emiliano, ai crimini del comunismo e dello stalinismo, a quella violenza politica che, ispirandosi alla contrapposizione tra fascismo e antifascismo, ha insanguinato il Paese negli anni di piombo. Anche oggi episodi di cronaca macchiano una identità nazionale che si riconosca in un passato condiviso. Mi vengono in mente gli insulti che accompagnano spesso, nel corteo del 25 aprile, la sfilata della brigata ebraica. *(Applausi)*. Ricordo le offese arrecate a Letizia Moratti, figlia di un partigiano, in passato costretta ad abbandonare, a Milano, il corteo del 25 aprile. Signor Presidente, voglio anche citare un episodio recente, che ha avuto luogo nella mia provincia. I vertici del Partito Democratico di Schio hanno festeggiato i cento anni di Valentino Bortoloso, detto Teppa, dichiarandosi onorati su Facebook di avergli stretto la mano e indicandolo come un protagonista della storia, con la "S" maiuscola. Peccato che Teppa si sia macchiato di un crimine orrendo, nel luglio 1945, quando, a guerra finita da oltre due mesi, insieme ad altri *ex* partigiani comunisti, irruppe nel carcere di Schio, massacrando 54 detenuti, alcuni dei quali fascisti, altri detenuti comuni, lasciando tante altre vittime ferite. Teppa ha concluso, insieme ai familiari delle vittime, un tortuoso percorso di riconciliazione, ispirato tra l'altro dal vescovo di Vicenza e oggi, espiata la sua pena, ha diritto di trascorrere in serenità gli ultimi anni di vita e non intendo certamente infierire contro di lui oggi. Ho criticato e critico anche oggi in quest'Aula l'operato dei dirigenti locali del PD, che hanno voluto celebrare addirittura pubblicamente su Facebook il suo compleanno, con dichiarazioni di encomio e di stima inaccettabili. Ho immediatamente invitato la segretaria del partito, Elly Schlein, a dissociarci da tale improvvida iniziativa. signor Presidente, ahimè il silenzio, per certi versi assordante. Ho invitato Giacomo Possamai, capogruppo in Regione Veneto del Partito Democratico, oggi candidato sindaco a Vicenza, la mia città, ma anche lui ha preferito soprassedere. rinnovo quindi l'invito anche oggi al Capogruppo Boccia, del Partito Democratico, a dissociarsi da quella iniziativa del tutto insensata *(Applausi)*, che rischia solo di avvelenare il clima locale. Mi sento di pronunciare questo invito con la serenità e la libertà intellettuale del figlio di un ragazzo che il 25 aprile aveva vent'anni e, in quel frangente, si trovava detenuto nel carcere di Bassano del Grappa, in quanto resistente antifascista cattolico (allora si diceva "partigiano bianco"). Mio padre, di quegli anni della sua giovinezza così difficili, mi ha trasmesso un ricordo sobrio, sempre tormentato, mai enfatico. Di fronte a quei drammi, vissuti dalla generazione dei nostri padri, credo ci si debba inchinare tutti oggi, indicando alle giovani generazioni, piuttosto distratte, una memoria il più possibile condivisa, basata sulla realtà storica.

Non posso negare di essere rimasto sorpreso dal fatto che il Partito Democratico e le altre opposizioni invece non voteranno quella di centrodestra, a prima firma del Se ho capito bene, vi disturbano i riferimenti al comunismo e alla caduta del Muro di Berlino, ma confesso di essere basito di fronte a questi argomenti. Capisco che con la svolta a sinistra imposta dalla nuova segretaria, ogni compromesso, anche il più ragionevole, con questa maggioranza sia divenuto impossibile, ma ne prendo atto. Mi sorprende anche la posizione di astensione del Terzo polo, perché gli argomenti che sono stati portati a conforto della loro posizione politica in realtà non mi hanno convinto, come prima ho detto. Rimane il rammarico per un'occasione perduta, signor Presidente, per avviarci ad una pacificazione e ad una memoria condivisa a cui entrambe le mozioni, almeno a parole, tendevano.

La libertà che questo luogo rappresenta, la libertà che strenuamente difendiamo, poggia sul sacrificio di molte vite umane, il sacrificio di donne e di uomini che hanno pagato il prezzo più alto, la loro stessa esistenza. Ebbene, ogni qualvolta noi mettiamo piede nel tempio della democrazia, abbiamo il dovere di ricordarcelo, come abbiamo il dovere di ricordarci di mettere in ogni nostra azione lo spirito che animò quelle battaglie. «Il fascismo è l'antitesi delle fedi politiche», disse il presidente Pertini. È forse oggi anacronistico ricordarlo. Io non credo, non lo è e non può esserlo fino a quando non cesseranno i tentativi di svuotare di significato queste parole

Presidente, perché chi rispetta la verità storica - e noi tutti abbiamo il dovere di rispettarla - fa da diga al disorientamento, alle apologie, ai pericolosi ritorni all'indietro. Sottacere o, peggio ancora, negare le sacche di negazionismo che si insinuano nella società e che, nell'ombra, minano la memoria comune, potrebbe essere un errore grave, che potrebbe costarci molto caro, Presidente. Ugualmente sarebbe un errore grave non accorgersene perché distratti dalle divisioni ideologiche. Quello che mi domando e le domando, Presidente, è se questo Governo e i suoi esponenti stanno facendo abbastanza per mantenere alta la guardia. Quello che invece so è che noi abbiamo la grandissima opportunità di ritrovarci coesi, come comunità, intorno a date simbolo per la nostra Nazione. Celebrare il 25 aprile, il 1° maggio o il 2 giugno non può essere un mero rito formale, quasi una prassi derubricata ad atto dovuto. Queste date sono un patrimonio immenso e lo sono per tutti gli italiani *(Applausi)*, indistintamente, di destra e di sinistra, cittadini di oggi e cittadini che verranno. In questo senso, il monito della senatrice Liliana Segre di vivere queste date con autentico spirito repubblicano non può andare disperso. Come lei stesso ebbe a dire, Presidente, il 25 aprile ci ricorda che resistere è necessario, è un dovere, oggi come allora. Le conquiste politiche e culturali che oggi ci appartengono, i diritti e le libertà di cui godiamo, sorgono quel giorno di settantotto E noi abbiamo il compito di essere degni custodi di questa eredità e di appellarci, oggi come allora, alla pace. Un'esigenza che travalica i confini nazionali e che, in questo momento, ci fa pensare naturalmente all'Ucraina. La *premier* Meloni ha dichiarato in quest'Aula che non ci sono le condizioni per la pace. signor Presidente, io non posso fare a meno di credere che non solo il momento della pace sia proprio questo, ma che il momento della pace sia sempre. Questo, inoltre, è anche il momento di garantire agli italiani un lavoro dignitoso sul piano morale, sociale ed economico; un lavoro che non contempli il rischio di rimetterci la vita, perché anche una sola morte è un evento è un evento inaccettabile. Questa è una sfida che non stiamo vincendo, dobbiamo dircelo chiaramente. Il 1° maggio rappresenta un baluardo per le istituzioni. È lì a ricordarci e a spronarci a fare meglio. Ora, onorare il fondamento della nostra civiltà, che è racchiuso nei principi della nostra Carta costituzionale, equivale innanzitutto a mobilitarci. Quindi, quale maniera migliore di partecipare attivamente ad una svolta sul piano dei diritti, che assicurare, come chiediamo da tempo, un salario minimo decoroso? Il 2 giugno, infine, celebra l'essenza della nostra Repubblica, i suoi principi fondativi, le sue istituzioni, le sue leggi, la sua organizzazione, ma non solo. Prendendo in prestito le parole del presidente Mattarella:, questa festa rappresenta la vita delle donne e degli uomini di questo nostro Paese, il contributo, grande o piccolo, che ciascuno di loro ha dato a questi decenni di storia comune. Come vedete, ognuna di queste date afferma la grandezza della nostra Patria; una grandezza che non dobbiamo dare per scontata, perché l'Italia è stata ricostruita dalle macerie e noi dobbiamo consegnarla, ai nostri figli e alle future generazioni, nella sua forma migliore: democratica, libera e giusta. Per tutti questi motivi, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla mozione n. 39, a prima firma del

l'invasione russa nei confronti dell'Ucraina ci ha riportato indietro nel tempo. Le scene di una guerra ripiombata nel nostro continente, le immagini di morte, di crudeltà, di orrore così vicine evidenziano, ancora una volta, quanto la pace sia un bene prezioso, da difendere ogni giorno, un bene fragile attaccato su diversi fronti quotidianamente. Quindi, è evidente la necessità di non abbassare la guardia quando la pace viene messa in discussione o semplicemente quando viene data per scontata. La nostra responsabilità, in quanto rappresentanti del popolo italiano, è proprio nel mettere in atto tutte le iniziative necessarie a custodire questo bene prezioso da consegnare alle future generazioni. E lo dobbiamo fare in modo coeso, in modo corale, dando esempio di unità di fronte ad un Paese che ci sta guardando. La mozione dell'opposizione riporta tratti del del discorso della senatrice Segre, pronunciato all'avvio dell'attuale legislatura, nella parte in cui dice che le grandi Nazioni dimostrano di essere tali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria. Perché non dovrebbe essere così per il popolo italiano? Perché mai dovrebbero essere vissute come date divisive, anziché con autentico spirito repubblicano, il 25 aprile, festa della liberazione, il 1° maggio, festa del lavoro, e il 2 giugno, festa della Repubblica? Anche su questo tema della piena condivisione delle feste nazionali, delle date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro, grande potrebbe essere il valore dell'esempio, di gesti nuovi e magari inattesi. Gesti nuovi e magari inattesi - lasciatemelo dire - che possono partire già oggi da quest'Aula. La mozione della maggioranza, invece, si richiama alla risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa e in particolare alla posizione unanime in essa espressa contro ogni potere totalitario, a prescindere da qualunque ideologia e segnatamente contro il nazismo, il fascismo e il comunismo. Occorre quindi riconoscere l'importanza delle date che ricordano momenti fondamentali della storia dell'Italia unita, libera e democratica, che non si limitano al 25 aprile, al 1° maggio, al 2 giugno, ma includono anche il 17 marzo, data della proclamazione del Regno d'Italia, il 4 il 4 novembre, Festa dell'unità d'Italia e delle Forze armate e altre date in memoria di pagine particolarmente significative, come il 27 gennaio, Giornata internazionale in memoria delle vittime della Shoah, il 10 febbraio, Giorno del ricordo in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il 18 aprile, quando gli elettori italiani collocarono la nostra Nazione nel mondo libero e democratico, e il 9 novembre, il Giorno della libertà quale ricorrenza dell'abbattimento del Muro di Berlino. impegno va quindi nel senso della necessità di richiedere la collaborazione di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche perché vengano adottate le opportune iniziative affinché le pubbliche commemorazioni di tutti gli avvenimenti della storia italiana ed europea si svolgano nel rispetto della dovuta accuratezza storica, senza trarne occasione per attacchi ad avversari che pure si riconoscono nei principi, nei valori e nel dettato costituzionale e affinché tali eventi rappresentino momenti di vera condivisione e partecipazione di tutte le componenti politiche e culturali che si riconoscono nei valori della libertà e della democrazia e rafforzano i sentimenti di unità nazionale, di inclusione, di perseguimento del bene comune e, ove necessario, di riconciliazione. conclusione, Presidente, a noi oggi l'onere di tradurre in atti concreti quanto troppo spesso rimane solo enunciato. La Lega lo farà votando convintamente a favore di entrambe le mozioni. l'opposizione a fare altrettanto, in un'ottica di reale conciliazione *(Applausi)*, ma dalle dichiarazioni che ho ascoltato questa è ancora molto distante dall'essere attuata. Noi siamo, sì, antifascisti e lo rivendichiamo, ma siamo anche contro i regimi comunisti e in generale contro tutti i sistemi totalitari, nessuno escluso e questa è la nostra differenza.

proprio quello di unire questa nostra Assemblea. Non a caso, è una mozione che non impegna il Governo, ma il Senato, e non a caso abbiamo voluto presentare le ragioni di questa mozione qui in quest'Aula, auspicando che nell'altro ramo del Parlamento questa discussione avvenga nei prossimi giorni, perché questa legislatura simbolicamente è iniziata qui, con le parole di Liliana Segre che hanno unito tutti noi e che hanno consentito a tutti noi

e se è vero che ci sono alcune date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro - cito sempre Liliana Segre e ricordo gli applausi di tutti noi - allora non capiamo perché, signor Presidente, l'Assemblea del Senato non possa impegnare se stessa per le commemorazioni delle date fondative della nostra storia, che è storia antifascista, che ha radici profonde, che è figlia di accadimenti che sono stati richiamati in quest'Aula e che noi abbiamo semplicemente il dovere di rinnovare per la memoria di tutti noi, per la memoria di chi verrà, dei nostri figli, per la memoria di queste mura, che ci accolgono ogni giorno e alle quali dobbiamo onore quotidiano. Signor Presidente, mi sarei aspettato un sostegno senza discussione, magari aprendo una discussione su cos'altro possiamo fare per il futuro, da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Intendo senza discussione sulla natura di quell'impegno, senatore Malan, che ha un'unica radice profonda: la radice antifascista della Repubblica Italiana *(Applausi)*, una radice che non abbiamo ritrovato nella mozione che non ci aspettavamo presentaste, ve lo dico con grande franchezza. Pensavamo infatti che le parole di Liliana Segre, che caratterizzano tre quarti della nostra mozione, e le parole del Presidente Mattarella, che rappresentano l'altro quarto della nostra mozione, fossero sufficienti fossero sufficienti *(Applausi)*. E invece no: quei quattro quarti non bastavano; era necessario provare ancora una volta a riscrivere. Colleghi, senza memoria non c'è futuro; la storia è una sola. La memoria dev'essere una ricostruzione condivisa dei fatti accaduti, un'elaborazione che si fa patrimonio comune che poi diventa lezione per il domani, ed evidentemente quella lezione non era bastata nel primo giorno di legislatura. L'antifascismo, cosa fu e che cos'è oggi, mi consentirete, visto che abbiamo due mozioni - non avrei fatto questo esercizio se ci fossimo ritrovati sulle parole della senatrice Segre e del presidente Mattarella fu una reazione morale e politica alla dottrina e alla prassi del fascismo al potere. Sorse soprattutto ad opera di alcune formazioni e partiti dell'Italia prefascista che disponevano della tribuna parlamentare e di una certa libertà di stampa; Dopo il delitto Matteotti, richiamato dai colleghi Verini e Verducci, votate le leggi dittatoriali del 1925, rivelatasi con la sconfitta dell'Aventino - l'impossibilità di un'efficace lotta antifascista sul piano della legalità e dentro le istituzioni, il fulcro della resistenza al fascismo passò all'estero,

e la concentrazione antifascista, sorta nel 1927 dall'unione di tutti gli antifascisti, comunisti e non comunisti, che erano, in un certo senso, la continuazione dell'Aventino. In Italia l'antifascismo restò retaggio dei gruppi operai che conservavano legami con il clandestino, perché diventò clandestino, come il presidente La Russia sa, il Partito Comunista, di non pochi aderenti, tanti aderenti - lo dico qui a chi vi si ispira del Partito Popolare e di un folto numero di intellettuali che ebbero come maggior rappresentante di riferimento Benedetto Croce. L'irrigidirsi del regime dittatoriale, il suo immiserirsi più in costrizioni anche formali, il volto imperialista del fascismo, la politica filotedesca, le aberrazioni razziste provocarono una crisi anche tra le diverse generazioni di allora. Si formò così in Italia quell'*humus* dal quale nacque la Resistenza, termine che alcuni estendono all'intero antifascismo, mentre altri lo riversano nella lotta clandestina tra il 1943 e il 1945. Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, l'antifascismo assunse in Italia le caratteristiche di un orientamento di cultura politica, che valorizza la Resistenza come momento fondante del nuovo patto costituzionale, esattamente il patto richiamato dalla senatrice Segre il primo giorno di legislatura e che oggi alcuni di voi rinnegano. Ecco perché la presidente Giorgia Meloni ha sbagliato a definire solamente «italiani» le vittime delle Fosse ardeatine, come se la guerra mondiale avesse visto gli italiani contro i tedeschi. No, c'erano gli antifascisti da una parte e i nazifascisti dall'altra con la complicità a volte involontaria, a volte drammaticamente inconsapevole, anche di alcuni cittadini italiani. Alle Fosse ardeatine furono uccisi barbaramente - come ha ricordato il senatore Verducci prima di me - 335 antifascisti, di cui 75 ebrei. Sì, colleghi, 75 ebrei, lo ricordiamo ogni volta: italiani ebrei. Questa è la verità storica. Fu un attentato di guerra quello di via Rasella, riconosciuto da sentenza negli anni Cinquanta, e il battaglione Bozen faceva parte dei reparti che rastrellarono Roma, formato da ufficiali tedeschi e soldati altoatesini. Non era una banda musicale; abbiamo apprezzato le scuse del presidente La Russa, perché sa come tutti noi che c'era una parte giusta e una parte sbagliata della storia e quei partigiani, onorevoli senatori, erano dalla parte giusta della storia. Il battaglione Bozen non solo non era una banda musicale, ma purtroppo era dalla parte sbagliata della storia. Se si applaude il discorso di Liliana Segre in Aula, come tutti abbiamo fatto, non si può dire che abbiamo che abbiamo fatto una valutazione diversa - lo dico col massimo rispetto per il collega Speranzon - sulle date che uniscono questo Paese, perché semplicemente si rischia di finire in un uso ideologico della storia. Chi non pronuncia mai la parola antifascismo, non solo non riconosce le radici della Repubblica, ma rischia di umiliarne la memoria. quello che vorremmo che accadesse in questi giorni che ci accompagnano al 25 aprile è che non ci fosse revisionismo, a volte involontario, a volte pensato, a volte ragionato, a volte anche reazionario che apra la strada all'indebolimento della democrazia e dei suoi pilastri, certamente della democrazia italiana. La memoria serve proprio a evitare che questo accada, perché se è vero che la libertà ha le sue stagioni e rischia di indebolirsi, noi abbiamo il dovere di nutrirla la libertà, di difenderla e viverla fino in fondo, di spiegarla ai ragazzi di oggi, di spiegare la genesi della nostra libertà, soprattutto in un campo caratterizzato da una da una mutazione capitalistica che è sotto gli occhi di tutti, da un mondo aperto e multietnico. In questo mondo non è possibile nessuna sostituzione etnica *(Applausi)*, perché è multietnico e lo sarà sempre più. Se qualcuno non l'ha capito, se lo faccia spiegare dai propri figli, perché sono in grado di spiegarcelo. Questa è la ragione di fondo per cui Resistenza e antifascismo democratico appaiono radici ancora più solide della nostra Repubblica ed è per questa ragione che ci aspettavamo un sostegno senza condizioni all'impegno che vi abbiamo chiesto.

Presidente, lo sforzo dei colleghi della maggioranza merita una motivazione chiara da parte del Gruppo Partito Democratico sul perché ci ritroviamo a non poter votare quella mozione e perché ci aspettavamo la condivisione della nostra del mio intervento, è la Festa della liberazione dal regime nazifascista, non è una ricorrenza comunista o estremista. Ci auguriamo che tutto il Parlamento della Repubblica italiana la sappia ricordare come il nostro Paese e la sua storia meritano. Il 1° maggio e il 2 giugno, indicati in quella

Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, colleghi dell'opposizione, evidentemente non ci avete visti arrivare *(Applausi)*, perché non avete capito che noi la votiamo la vostra mozione, perché

peraltro, non è necessario ripeterle, altrimenti potevamo copiarla e presentarne un'altra e un'altra ancora. Potevamo benissimo farlo. Noi vorremmo - ed è il nostro auspicio per adesso e per il futuro che il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e le altre date che abbiamo inserito nella nostra mozione, di cui parlerò, fossero veramente un momento di condivisione.

manifestazioni del 25 aprile e alle altre manifestazioni. Non hanno dato un buon esempio coloro che alle manifestazioni del 25 aprile hanno fischiato e spintonato gli eroi della brigata ebraica e su questo non ho mai sentito forti dissociazioni. *(Applausi).* Oggi poteva essere l'occasione per dire: 25 aprile inclusivo anche per la brigata ebraica. *(Applausi).* perché nell'esercito britannico hanno partecipato a quella guerra che ha portato al 25 aprile. Visto che voi dite che noi dovevamo aggiungere quella parola, devo dire che il più esplicito è stato il senatore Boccia: noi non dovevamo presentare nulla, questo nell'ambito di un pluralismo democratico. Loro scrivono, non ci consultano e dobbiamo votare senza discussione. Poi si è detto che possiamo anche parlare e dire quanto è bella la mozione e infatti la votiamo.

per il 25 aprile è stata spintonata in nome dell'antifascismo *(Applausi)*, lei che è figlia di un partigiano e, peraltro, rappresentante delle istituzioni.

siamo stati graditi, però, ai cittadini italiani che ci hanno dato la maggioranza in Parlamento grazie alla nostra Costituzione. Veniamo proprio alla Costituzione. Stando al criterio

che noi ci richiamiamo alla risoluzione del Parlamento europeo, che condividiamo, in cui si condannano tutti i regimi totalitari, a prescindere dalle ideologie, come il nazismo, il fascismo e il comunismo. Allora essere contro il fascismo non è essere così? Senatore Magni, la prego. magari ha avuto colleghi di partito che hanno avuto l'urgenza di andare altrove in quel momento *(Applausi)*, perché cita alcuni fatti che si potevano anche aggiungere. Per esempio, cita il 23 agosto 1939 come data da ricordare, perché ha compromesso la libertà di interi popoli europei a causa dell'accordo della Russia di Stalin con la Germania di Hitler *(Applausi)*, cosa che - nell'ambito di una memoria che si vorrebbe condivisa - è stata a lungo nascosta dalla storiografia, in particolare nei libri di testo. Allora, stando al vostro criterio, chi era nell'Assemblea costituente non avrebbe dovuto votare la Costituzione, perché nella Costituzione la parola antifascista non c'è.

Purtroppo è una mentalità, è quello che diceva il senatore Speranzon, citando Ernesto Galli della Loggia, cioè che un certo antifascismo ha fatto allontanare da questa forma di manifestazione antifascista coloro che, se solo si discostano appena da ciò che vuole qualcuno, che ha la verità in tasca, nell'esprimere il proprio sostegno alla nostra Costituzione,

in questo contesto abbiamo pensato di aggiungere alle date - che abbiamo compreso con le stesse parole che avete usato voi - delle altre date. Il 25 aprile è una data fondamentale per la nostra democrazia, perché se non fosse stato sconfitto il regime fascista, non sarebbero arrivati la Costituzione, la Repubblica, la democrazia e le libere elezioni. Se però il 18 aprile 1948 gli elettori italiani non avessero collocato l'Italia nel campo delle democrazie, che si riconoscono nei valori della democrazia, della libertà e dei diritti individuali, la libertà non ci sarebbe stata e ci sarebbe stato un altro tipo di dittatura. per chi dice che il comunismo non ci interessa, perché non ha toccato Qualcuno dice che il comunismo non ci interessa, perché non ha toccato l'Italia. I 10.000 morti - non meno - delle foibe e degli altri massacri delle minoranze giuliano-dalmate furono causati dai partigiani comunisti di Tito. Allora non è vero che il comunismo non l'ha toccata. In secondo luogo, il comunismo non ha toccato l'Italia grazie al voto degli elettori il 18 aprile 1948 In terzo luogo, a coloro che hanno l'Europa sempre sulle labbra ricordo che l'Europa non finisce ai nostri amatissimi confini, ma si estende a tanti Paesi europei che hanno subito gravissime dittature comuniste. Aggiungo una cosa, per fare una precisazione: la Costituzione fu approvata anche con l'apporto del Partito Comunista. I partigiani comunisti ebbero un ruolo importantissimo nella Resistenza... *(Commenti)*, ma c'erano anche altre ma c'erano anche altre formazioni, che si è sempre un po' ignorato, così come si sono ignorati a lungo gli internati militari in Germania, così come si sono ignorati a lungo coloro che hanno combattuto nell'esercito italiano regolare, fedele al suo giuramento al re. Pertanto, c'è stata una certa scelta nel commemorare, mentre bisognerebbe essere inclusivi. fare di queste date un patrimonio comune. Come dicevo, la Costituzione ha avuto un grosso contributo da parte del Partito Comunista, guidato da quel Palmiro Togliatti, grande politico, che ha avuto la maturità

siamo a favore di tutto, della vostra mozione, della celebrazione della fine del totalitarismo, qualunque esso sia, in quel caso il totalitarismo fascista, ma riteniamo che si debba essere ben coscienti del fatto che non vogliamo vivere in un eterno 1944. Noi siamo per il 1945, la fine della guerra, per il 1946, il 1947 e il 1948, in cui si scrisse la Costituzione e anche anche coloro che non parteciparono alla scrittura della Costituzione poterono partecipare alle elezioni del 1948, a tre anni dalle gravissime... prego di avviarsi a concludere, difendendo gelosamente e strenuamente tutte le libertà che la nostra Costituzione garantisce e incarna.

nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per lo sport e i giovani.

Nel comunicato finale si riafferma l'impegno del G7 e dell'Unione europea ad affrontare le sfide globali, inclusi il cambiamento climatico, la salute, la sicurezza alimentare ed energetica e la migrazione irregolare. Si afferma l'impegno a sostenere e rafforzare l'ordine internazionale libero e aperto, basato sullo stato di diritto; a promuovere una pace comprensiva giusta e durevole in Ucraina, in linea con quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Si riafferma l'impegno a rafforzare la cooperazione con i *partner* nell'Indo- Pacifico, in Medio Oriente, in Africa, in Asia Centrale, America Latina e Caraibi. L'aggressione russa all'Ucraina continua a richiedere un costante impegno del G7 su molteplici fronti, ad esempio nel sostegno alla resilienza ucraina, nella promozione di una soluzione pacifica del conflitto in linea con la risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nonché nella futura ricostruzione del Paese. L'importanza del continente africano, relativamente al quale l'Italia ha guidato la discussione, e la gravità della crisi in corso in Sudan ed in Tunisia fanno emergere l'esigenza, per il G7, di assumere un ruolo maggiormente incisivo nelle questioni legate allo sviluppo del continente, rafforzando la collaborazione con l'Africa. È necessario anche preservare il carattere libero ed aperto dell'Indo-Pacifico, agendo insieme all'ASEAN e agli altri *partner* nella regione secondo principi condivisi, improntati alla risoluzione pacifica delle dispute nonché alla tutela dell'integrità territoriale delle libertà fondamentali e dei diritti umani. Le chiedo quindi, ministro Tajani, quali siano gli esiti della predetta riunione e quali iniziative abbia intenzione di intraprendere per favorire un rafforzamento del partenariato G7-Africa e della collaborazione con i Paesi asiatici, continuando ad assicurare nell'agenda del G7 la centralità del continente africano e dell'Indo-Pacifico nei processi decisionali relativi alle sfide globali, anche in vista della Presidenza italiana del 2024.

e Sudan lo impongono. Ma non possiamo limitarci a inseguire le emergenze: l'Africa deve essere una priorità della nostra azione di politica estera anche per quanto riguarda le sfide trasversali e di lungo periodo, quindi quella della migrazione irregolare. Ho riaffermato per questo la necessità che il G7 rilanci il partenariato con l'Africa e assuma un ruolo di primo piano nelle questioni riguardanti sviluppo, lotta ai cambiamenti climatici, salute, sicurezza alimentare, migrazioni regolari e infrastrutture. Dobbiamo adottare un'azione strategica di diplomazia per la crescita secondo le stesse linee che ispirano l'approccio italiano del piano Mattei. In stretto rapporto con la Presidenza giapponese e con gli Stati Uniti ho inoltre promosso l'organizzazione di una riunione straordinaria del G7 sul Mediterraneo e sul Medio Oriente, possibilmente in formato allargato ai Paesi della Regione. Sottolineata questa priorità politica, discuteremo ora modalità e risultati attesi per questo G7 *plus*, il cui obiettivo è la stabilizzazione di un'area cruciale per gli equilibri globali. La riunione dei Ministri degli esteri del G7 ha dedicato forte attenzione anche all'Indo-Pacifico. Ho assicurato la volontà dell'Italia di assumere un ruolo ancora più visibile e attivo in linea con i crescenti interessi nazionali nella regione. La nostra è una strategia a tutto campo che abbraccia gli aspetti politici, di sicurezza ed economici. La campagna del pattugliatore polivalente d'altura Morosini appena avviata durerà cinque mesi e comprenderà anche esercitazioni congiunte con le marine dei Paesi alleati e amici, a testimonianza dell'attenzione per il tema delicato della sicurezza marittima e del rispetto del diritto internazionale del mare. L'anno prossimo a essere impegnata nella regione sarà la nave scuola Vespucci. toccherà dodici Paesi, tutti di crescente interesse dal punto di vista industriale e parteciperà ad alcuni dei più importanti eventi fieristici nel settore della difesa. Il rafforzamento dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano in tutti i comparti di punta e il sostegno alla già estesa

altrettanto importanti e vogliamo rendere l'Italia protagonista anche in queste aree strategiche sul piano geopolitico ed economico. ringrazio, ministro Tajani, per la sua risposta, di cui sono molto soddisfatto, perché oltre a essere stata precisa e puntuale, è in linea con i principi che hanno sempre ispirato l'azione di Forza Italia e del centrodestra in politica estera. Ha parlato di pace, di cooperazione, di libertà, di ricostruzione, di diritti, di diplomazia, di piano Mattei, di sicurezza, di valori comuni. Le sue parole non possono che rassicurare noi parlamentari e tutti gli italiani. La ringrazio per il lavoro che svolge quotidianamente, che consente al nostro Paese di tornare ad avere una politica estera chiara

La ringrazio per il lavoro che svolge quotidianamente, che consente al nostro Paese di tornare ad avere una politica estera chiara e incisiva, che riporta finalmente l'Italia a essere protagonista dello scenario internazionale, donandole quella centralità che merita. Buon lavoro, ministro Tajani.

ripercorriamo insieme la vicenda della vendita di bombe italiane agli Emirati che - come lei sa - è stata bloccata dai Governi Conte 1 e 2, in considerazione del loro utilizzo contro la popolazione civile yemenita, e sbloccata da questo Governo per motivazioni di cui oggi le chiediamo spiegazione. A fine luglio 2019, il Governo Conte 1 - come lei sa - anche a seguito dell'approvazione di una nostra risoluzione alla Camera, decideva la sospensione, per diciotto mesi, delle licenze di esportazione di bombe aeree e missili verso gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, e introduceva la richiesta di un certificato di utilizzo finale rafforzato su tutte le altre forniture militari. A fine gennaio 2021, il Governo Conte - a seguito dell'approvazione di una risoluzione del MoVimento 5 Stelle in Commissione esteri - decretava la revoca definitiva delle vecchie licenze di esportazione di bombe aeree e missili verso gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, confermando la sospensione di future licenze analoghe. Arriviamo ad oggi, Ministro. Il 17 aprile 2023, l'altro giorno, questo Governo decreta la libera esportazione di materiale d'armamento verso gli Emirati Arabi Uniti, rimuovendo anche il blocco all'*export* di bombe aeree e missili, bloccato dal 2019. Il Governo lo fa spiegando che le forniture militari ad Abu Dhabi non ricadono più tra i divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, che disciplina il commercio di armi. Ma tale condizione, Ministro, a nostro giudizio non corrisponde al vero. Infatti, se è vero che la citata legge n. 185 vieta la vendita a Paesi in guerra, è altrettanto vero che la guerra in Yemen, seppure in tregua, non è ancora terminata con un accordo di pace. Inoltre, l'impegno militare degli Emirati Arabi Uniti nel Paese yemenita non è affatto terminato, come dimostra la perdurante occupazione illegale della strategica isola yemenita di Socotra, dove le forze d'occupazione intendono stabilire militarmente la loro permanenza. Ministro, in definitiva, continuano ancora oggi a permanere tutte le condizioni previste dalla legge n. 185 perché l'Italia conservi il diritto di esportazione di armi e, alla luce di tutto quanto esposto, chiediamo a lei di darci delle spiegazioni.

L'Italia ha aderito - fin dall'inizio del conflitto in Yemen - all'embargo sulla vendita di armi decretato dall'ONU nei confronti dei ribelli Houthi. Tale embargo non si estendeva ai Paesi della coalizione intervenuta a sostegno del legittimo Governo yemenita. Le esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, pur soggette a un attento scrutinio, non sono mai state interrotte dall'Italia e dalla maggioranza dei Paesi dell'Unione europea. Nel 2021, l'Italia ha concesso licenze verso gli Emirati per un valore di 56 milioni di euro, la Germania per 36 milioni, la Spagna per 120 milioni, la Svezia per 864 milioni e la Francia per oltre 16 miliardi. L'Italia ha sospeso - nel luglio 2019 - a seguito di un atto di indirizzo parlamentare, le vendite verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi di alcune tipologie di armi che potevano essere utilizzate contro la popolazione civile in Yemen. Una revisione di queste misure restrittive verso gli Emirati è stata decisa nell'agosto del 2021 dal Governo allora in carica, anche sulla base di un atto del Parlamento in tal senso. La decisione presa lunedì dal Consiglio dei ministri conferma e rafforza, quindi, una misura già da tempo in vigore. Nel corso del 2022 e del 2023 la situazione in Yemen è sensibilmente migliorata. Dall'aprile dello scorso anno le attività militari sul terreno sono limitate; la tregua ha di fatto tenuto. Sul terreno non si è verificata una ripresa delle ostilità, al di là di scontri episodici. Negli ultimi giorni l'attività diplomatica ha registrato un'accelerazione; le parti hanno scambiato circa 900 prigionieri: è un segnale importante per la ripresa del processo politico. Di questi sviluppi ha dato atto, a più riprese, l'inviato speciale per lo Yemen del segretario generale delle Nazioni Unite Grundberg: al Consiglio di sicurezza ONU ha riferito che i livelli di violenza del conflitto restano bassi e che esistono tutti i presupposti per una cessazione duratura e strutturata delle ostilità. La notevole diminuzione delle operazioni belliche sta riducendo significativamente il rischio di uso improprio di armi, in particolare contro obiettivi civili. Gli Emirati, dopo aver annunciato il ritiro dalle operazioni militari in Yemen, hanno sostenuto gli sforzi diplomatici della coalizione, con Riad in testa, per dialogare con gli Houthi e porre fine al conflitto. Nel 2022 hanno confermato il loro significativo contributo finanziario per la stabilizzazione e la ricostruzione del Paese. Anche il riavvicinamento tra Riad e Teheran potrà ora produrre effetti positivi sulla situazione in Yemen, rafforzando le condizioni per la pace. Prendendo atto dei progressi descritti, il Consiglio dei ministri ha voluto esprimere una chiara volontà politica di rilanciare le relazioni bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti a tutti i livelli. I miei colleghi del G7, che ho appena incontrato in Giappone, hanno salutato con favore questa nostra decisione. Il comunicato finale della riunione dei Ministri degli esteri del G7, che abbiamo approvato, ha espresso apprezzamento nei confronti del Governo yemenita, degli Emirati Arabi Uniti, oltre che dell'Arabia Saudita e dell'Oman, proprio perché si è raggiunta una situazione completamente differente. Quindi, c'è un riconoscimento unanime dai Paesi del G7 dei grandi progressi che sono stati fatti

più di un anno fa, aveva approvato una dura risoluzione di condanna del Governo emiratino per la sistematica persecuzione dei difensori dei diritti umani e per l'intensificazione della repressione della libertà di associazione, riunione ed espressione.

tali armi. Crediamo effettivamente che questo Governo sia supino, quasi ossessionato dalla corsa al riarmo, verso questi interessi delle *lobby* dell'industria. Non è un mistero che il Ministro della difesa sia un ex lobbista del settore delle armi. *(Applausi)*. Noi riteniamo che queste circostanze siano offuscando la lucidità

2023, Artem Uss, l'imprenditore russo figlio del governatore della regione di Krasnojarsk ed esponente politico del partito "Russia unita", è evaso dagli arresti domiciliari a Basiglio, nel sud di Milano; Era ai domiciliari a seguito di una decisione della magistratura sulla base di un mandato di cattura emesso negli Stati Uniti per l'accusa di numerosi reati, tra cui la violazione dell'embargo nei confronti del Venezuela, il contrabbando di petrolio, frode bancaria, riciclaggio e soprattutto contrabbando di tecnologie militari dagli Stati Uniti verso la Russia. Secondo quanto ricostruito dagli organi di stampa, in data 11 novembre gli Stati Uniti hanno avanzato la richiesta di estradizione e il 19 ottobre, due giorni dopo il fermo, il procuratore di New York aveva inviato al Ministro della giustizia una nota con la quale si avvertiva «dell'altissimo pericolo di fuga del detenuto». Il 25 novembre la corte d'appello di Milano ha stabilito gli arresti domiciliari e, a seguito di tale decisione, le autorità statunitense hanno inviato una nuova nota al Governo, evidenziando, dato l'altissimo rischio di fuga che Uss presenta, quanto virgolettato: «esortiamo le autorità italiane a prendere tutte le misure possibili per disporre, nei confronti di Uss, la misura della custodia cautelare per l'intera durata del processo di estradizione». La nota con la quale il Dipartimento di giustizia statunitense chiedeva all'Italia di non concedere i domiciliari, visto l'alto rischio di fuga, sarebbe stata inviata al Ministero della giustizia in data 29 novembre. Tuttavia, tale nota sarebbe stata inoltrata alla corte d'appello di Milano solo il 19 dicembre, dunque venti giorni dopo la sua ricezione. Al di là degli aspetti di carattere tecnico, su cui il ministro Nordio risponderà in altra sede, a noi in questa sede, signor Ministro, preme sottolineare come la fuga di Artem Uss, un uomo politico molto vicino al presidente Vladimir Putin, mini la credibilità dell'Italia di fronte a un alleato storico quale gli Stati Uniti, oltre che all'intera comunità internazionale, vista la particolare congiuntura che il nostro Paese e i Paesi *partner* stanno vivendo a seguito del conflitto ucraino. Vogliamo quindi sapere da lei qual è la sua valutazione in ordine alla credibilità del nostro Paese nei rapporti con gli Stati Uniti e in generale di fronte all'intera comunità internazionale per questo evento che si è consumato sul nostro territorio nazionale.

Signor Presidente, l'evasione dell'imprenditore russo Artem Uss è un fatto grave, su cui è importante fare piena chiarezza. Come ha appena riferito il ministro Nordio alla Camera, la decisione della corte di appello di Milano sull'applicazione degli arresti domiciliari al detenuto rientrava nell'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. Il Governo non aveva potere di intervento, né sulla sostituzione della detenzione con gli arresti domiciliari, né sull'impugnazione del provvedimento. Il ministro Nordio ha sottolineato che la procedura applicabile al caso non poteva essere quella prevista dall'articolo 714 del codice di procedura penale, menzionato dagli interroganti. Questa norma conferisce, infatti, al Ministro della giustizia la facoltà di richiedere misure coercitive, ma solo nel caso in cui all'atto dell'arresto sia già pendente una richiesta di estradizione. Al momento dell'arresto di Artem Uss, il 17 ottobre 2022, non pendeva alcuna domanda di estradizione. Il Governo ha quindi correttamente applicato l'articolo 716 del codice procedura penale, che prevede la revoca dell'arresto qualora il Ministro della giustizia non chieda entro dieci giorni il mantenimento della custodia in carcere; richiesta che il ministro Nordio ha trasmesso alla corte d'appello di Milano il 20 ottobre 2022. Il Ministro non aveva facoltà di intervenire nei seguiti della procedura. Riguardo alla nota richiamata dagli interroganti, con cui il Dipartimento di giustizia americano evidenziava l'alto rischio di fuga del detenuto, il ministro Nordio ha precisato che che essa non conteneva alcun elemento di novità rispetto a quanto già comunicato da Washington il 19 ottobre 2022 e condiviso con l'autorità giudiziaria il giorno dopo. Essa tuttavia è stata inviata alla corte d'appello di Milano il 23 dicembre 2022. Non è corretta, infine, la ricostruzione secondo cui la richiesta di sequestro dei dispositivi in possesso di Artem Uss sarebbe stata avanzata da parte americana dopo aver saputo della concessione degli arresti domiciliari. Essa risale, invece, al 15 ottobre 2022 ed era contenuta nella richiesta di arresto. Nei verbali non è presente, tuttavia, alcun riferimento ai dispositivi elettronici nella disponibilità di Uss, né al momento dell'arresto, né a quello della sottoposizione agli arresti domiciliari, eseguita il 2 dicembre 2022. Anche nel caso fossero stati rinvenuti nella procedura applicabile, quella appunto dell'articolo 716 e non dell'articolo 714 del codice di procedura penale, il sequestro è comunque obbligatorio e il Ministro della giustizia non ha potere di verifica *ex post.* Ciò premesso, alla luce della gravità di quanto accaduto, il Ministro della giustizia ha avviato azione disciplinare nei confronti dei componenti della corte di appello di Milano che hanno affievolito la misura cautelare verso Uss, in difetto di adeguata valutazione del rischio di fuga. Nei nostri continui contatti con gli Stati Uniti abbiamo confermato l'impegno delle autorità italiane nelle attività di indagini in corso. Abbiamo assicurato la la disponibilità a condividere tempestivamente con Washington ogni informazione attraverso i canali bilaterali più appropriati, mentre stiamo verificando l'attivazione della procedura di congelamento dei beni del signor Uss in Italia. America ed Europa sono le stelle polari della nostra politica estera. Il rapporto con gli Stati Uniti è e continuerà a essere solido e leale; così come incondizionato è il sostegno del Governo all'Ucraina, che troverà ulteriore conferma con la Conferenza per la ricostruzione in programma a Roma il 26 aprile. Concludo dicendo che è un impegno unanimemente riconosciuto e apprezzato dai nostri *partner*, a cominciare dagli Stati Uniti, come ribadito dal segretario di Stato americano Blinken nei numerosi colloqui che abbiamo avuto in occasione del G7 appena concluso in Giappone.

di queste parole e lo diciamo con grande rispetto della sua funzione, oltre che della sua persona. Ci saremmo attesi che in quest'Aula parlasse il Ministro degli affari esteri e che lei non si trasformasse in un portavoce del Ministro della giustizia. Lo abbiamo ribadito in altre circostanze e in altre occasioni. In questi minuti i nostri colleghi alla Camera stanno interrogando il ministro Nordio. Qui il punto, signor Ministro, non è tanto trincerarsi dietro una burocratica e difensiva interpretazione di normative, codicilli e procedure, quanto il fatto che in quella lettera che il Dipartimento di Stato ha inviato al Governo della Repubblica italiana venivano citati addirittura sei casi nei quali detenuti sottoposti a procedimenti di estradizione nel nostro Paese non sono stati tradotti conseguentemente. In altre parole, detta in maniera più volgare, l'Italia si è fatta scappare sei volte persone che dovevano essere estradate. E in quel contesto i nostri alleati ci dicevano di fare attenzione perché questo caso poteva diventare il settimo e così è stato. Abbiamo visto una fiera dello scaricabarile sulla vicenda che non si vedeva più in questo Paese dai tempi dell'evasione di Kappler. Di fronte a tutto questo, anziché risponderci dal punto di vista della capacità di un'assunzione di responsabilità, si viene sostanzialmente a dire che il problema è del ministro Nordio, che lo scarica sulla magistratura. In tutto questo la lettura che viene fatta dall'esterno dell'Italia è evidentemente purtroppo un grado di inaffidabilità delle istituzioni del nostro Paese, che viene ancora confermata dall'insufficienza di una risposta emanata e portata in questa sede. finestra"). La Presidenza ringrazia comunque il ministro Tajani per avere dato una risposta su un argomento che non è di sua stretta competenza. Grazie, signor Ministro.

crisi climatica, di salvare l'ambiente e il futuro dello sci. La preoccupazione è quindi forte anche tra gli addetti ai lavori, perché gli effetti del cambiamento climatico stanno avendo ripercussioni sugli stessi sport invernali. Eventi come la crisi siccitosa stanno colpendo anche questo mondo e, quando diciamo che il contrasto ai cambiamenti climatici non è più rimandabile, significa che dobbiamo agire adesso. Per questo motivo torno oggi a parlare in quest'Aula con lei, ministro Abodi, dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 e, in particolare, della pista da bob che verrà realizzata a Cortina, per appellarmi al suo buonsenso. La testardaggine con la quale si intende portare a compimento questa opera faraonica, nonostante i dubbi iniziali da parte del CIO; nonostante il forte impatto economico dell'opera, stimato in 120 milioni di euro; nonostante il forte impatto ambientale, sta superando ogni ragionevole limite. In questa sede vorrei soffermarmi sulle criticità che la realizzazione della pista da bob provocherà alle risorse idriche del territorio ampezzano, sapendo che la siccità siccità non ha lasciato indenni neanche le Dolomiti. La carenza d'acqua sta provocando grandi difficoltà anche nella provincia di Belluno, dove ARPA Veneto, nel suo rapporto del 31 gennaio 2023, parla di situazione grave, a causa di precipitazioni al di sotto della media storica e della scarsa presenza di neve. È un quadro preoccupante, in una provincia servita da un acquedotto in pessime condizioni che - come noto -perde a destinazione circa il 70 per cento dell'acqua captata dalle sorgenti. È sconcertante che si sia deciso di rifornire la pista da bob prelevando oltre 3.000 metri cubi di acqua dell'acquedotto comunale, sottraendo questa importante quota di risorse idriche alla comunità del territorio, sapendo peraltro che l'acquedotto comunale risulta già risentire della grande presenza turistica. Il rifacimento della pista da bob a Cortina causerà inoltre la deforestazione di un'area stimata di 20.000 metri quadrati, con l'abbattimento di 200 larici storici. Per questo mi rivolgo a lei, signor Ministro, per chiedere come intenda il Governo affrontare la vicenda e garantire al contempo che l'enorme consumo di acqua, necessario al funzionamento della pista da bob di Cortina, non comprometta le risorse idriche al servizio dei cittadini nel Comune di Cortina e, più nel dettaglio, se questo argomento verrà affrontato dalle autorità individuate di recente nel cosiddetto decreto siccità, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.

Innanzitutto, è opportuno segnalare che l'intervento di riqualificazione della pista "Eugenio Monti", adibita alla disciplina del bob e parabob, slittino e *skeleton*, è stato approvato a seguito dei positivi esiti della conferenza dei servizi decisoria sincrona indetta sul progetto definitivo della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, il 18 gennaio 2023. Per quanto riguarda l'asserito impoverimento del suolo e il rischio di permeabilità del terreno, a seguito della deforestazione, si segnala che all'interno della documentazione progettuale approvata in occasione della suddetta Conferenza dei servizi è presente una specifica relazione di riduzione forestale, concordata e approvata dall'ente preposto al rilascio delle relative autorizzazioni. È quindi opportuno segnalare che l'intervento prevede un progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di opere a verde di riforestazione dell'area e rimboschimento compensativo, nonché il versamento sull'apposito fondo regionale di un importo ricompreso all'interno del quadro economico dell'intervento, per il miglioramento colturale di una superficie doppia rispetto a quella di cui è stata richiesta la riduzione forestale e che sarà a disposizione dell'ente per specifiche opere di compensazione. Per quanto attiene al prelievo di acqua dal torrente Boite, tale soluzione è stata scartata nel corso della progettazione dell'intervento, non tanto per la limitata portata idrica - come da lei riferito - quanto per una precisa scelta di riduzione degli impatti dell'intervento sulle matrici ambientali, come peraltro illustrato nel corso della conferenza dei servizi decisoria, indetta dalla società Infrastrutture Milano Cortina per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento. Sono state infatti presentate, in quella occasione, le soluzioni tecnologiche alternative individuate per l'alimentazione dell'impianto di refrigerazione della pista, che non comportano prelievo di acqua dal Boite. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse idriche, già in sede di conferenze dei servizi è emersa la necessità di coniugare il necessario accumulo idrico richiesto per il funzionamento della nuova infrastrutture sportiva, con l'attualmente limitata disponibilità di risorse idriche prelevabile dalla rete del servizio idrico integrato. Il fabbisogno idrico complessivo, per garantire i consumi legati alle attività di carattere agonistico sportive, ai servizi igienico-sanitari previsti e ai consumi tecnici legati al mantenimento della refrigerazione della pista, è stimato in 21.000 metri cubi l'anno. Al fine di individuare la soluzione più idonea per risolvere tale criticità, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ha promosso la stipula di una convenzione con le seguenti amministrazioni ed enti competenti, già coinvolte nella conferenza dei servizi: Bim gestione servizi pubblici, Spa gestore nell'ambito del servizio idrico integrato; Consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi", ente di governo nell'ambito territoriale ottimale dell'Alto Veneto, e il Comune di Cortina d'Ampezzo. La soluzione individuata prevede la sostituzione di un vetusto serbatoio di compensazioni, localizzato in località Cadin, che attualmente non garantisce un adeguato accumulo per le ulteriori esigenze eccedenti le attuali utenze, e la necessità di un adeguamento tecnico infrastrutturale. L'accumulo idrico, così rinnovato, avrà un volume di circa 1.000 metri cubi e una capacità che consentirà di aumentare significativamente l'accumulo idrico, garantendo sia la copertura di picchi di consumo ben maggiori di quanto oggi possibile, sia la disponibilità idrica in fase di preparazione e avvio stagionale della pista refrigerata. Gli importi connessi alla realizzazione di tale infrastruttura, stimati in 2 milioni di euro, sono ricompresi all'interno delle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento di riqualificazione della pista «Eugenio Monti». in chiusura, il gestore d'ambito del servizio idrico integrato ha manifestato ampia disponibilità a realizzare gli interventi in oggetto di ampliamento del serbatoio idrico, ai sensi della suddetta convenzione, in ottemperanza agli interventi connaturati con la gestione d'ambito affidata. Il consiglio di bacino "Dolomiti Bellunesi" ha confermato l'intendimento di favorire il potenziamento del servizio idrico integrato, promuovendo la sinergia anche con altri soggetti pubblici che possono affiancare la realizzazione degli interventi già programmati a carico della predisposizione tariffaria. Il Comune ha condiviso la realizzazione dell'opera di potenziamento del servizio idrico integrato sul proprio territorio, impegnandosi a favorire le soluzioni anche amministrative correlate. La società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 ha confermato di poter fattivamente assolvere ai propri compiti istituzionali, anche in collaborazione con i soggetti pubblici locali, al fine di adeguare le infrastrutture del territorio collegate alle opere olimpiche. La realizzazione del nuovo serbatoio potrà così mettere al servizio dell'intera collettività locale la maggior capacità di stoccaggio idropotabile realizzata, oltre che garantire le esigenze di approvvigionamento idrico dell'impianto sportivo senza dover dedicare una specifica infrastruttura in una logica di sistema territoriale. In aggiunta a quanto precedentemente esposto, si segnala infine come riscontrabili dagli atti della suddetta Conferenza dei servizi che sono state previste, nell'ambito del progetto di riqualificazione della pista «Eugenio Monti», tutte le necessarie misure di tutela finalizzate ad una riduzione dei rischi di impatto ambientale delle lavorazioni e previsti i piani di monitoraggio ambientale sulle matrici maggiormente sensibili del rumore e dell'atmosfera. Il progetto della nuova pista di Cortina, così come tutte le opere contenute nel piano degli interventi, resta e resterà oggetto dei lavori della cabina di regia voluta dal Governo, che si riunisce ormai regolarmente ogni quindici

a seguire tutto il territorio ampezzano. Concorderà con me che costruire un serbatoio in una fase così siccitosa, in cui ogni goccia è preziosa, non vuol dire che si riempie di acqua. Da ex atleta ed ex sportiva ambientalista, so che la passione per lo sport e i valori può essere conciliata con la sostenibilità ambientale. Non servono quindi solo parole o la carta: servono delle azioni concrete che lei non ha saputo dirmi in questo momento. Non chiedo neanche di avere il coraggio di prendere decisioni forti. Chiedo di osare per essere faro anche rispetto a un contesto internazionale che potrà seguire il nostro esempio. Quindi, oltre a chiedere di ascoltare di nuovo le istanze dei comitati che sono tremendamente preoccupati in questo senso, anche per le conseguenze del contrasto del cambiamento climatico, a questo punto chiedo, anche a nome degli atleti e delle atlete di questa e delle future

gentile ministro Abodi, nel giorno in cui 13 milioni di tifosi sono in attesa finalmente di una parola di verità da parte della corte federale di appello nei confronti della squadra della Juventus, con la collega Sbrollini ho pensato di interrogarla sui casi di discriminazione nello sport. Tra il 2021 ed il 2022 l'Osservatorio nazionale contro le discriminazioni nello sport ha documentato 211 casi di discriminazione e violenza, una media di sedici al mese. Abbiamo tutti ben fissi nella memoria gli ultimi gravissimi episodi di violenza negli stadi, da ultimo gli scontri allo stadio Maradona durante Napoli-Milan lo scorso 2 aprile. Lei, signor Ministro, più volte, anche negli ultimi giorni, ha richiamato la necessità di un'azione comune e condivisa, anche con le società sportive, per debellare tali fenomeni alla radice, promuovendo una cultura dello sport che ne rispecchi i valori più nobili: la solidarietà, il *fair play*, il rispetto degli avversari, che nemici non sono da battere, ma semplicemente *competitor* con cui condividere una passione. Ciò che chiediamo al Governo e a lei, signor Ministro, è cosa intenda fare il Governo, nel breve e lungo periodo, per risolvere definitivamente questa che sta assumendo i tratti di una vera emergenza, magari prendendo spunto dai successi della Gran Bretagna. Servono certamente misure punitive, anche più severe del Daspo. Ma, insieme ad esse, è fondamentale avviare un grande lavoro culturale

giovani*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio per il quesito sottoposto alla mia attenzione, perché mi offre una occasione particolare non solo di confronto e di riflessione, ma anche per informare il Parlamento, doverosamente, sulle iniziative che, come Governo, stiamo ponendo in essere, per finalizzare tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto alle discriminazioni e al razzismo, con riferimento sia a quelle individuali che collettive. Voi sapete che io più volte ho cercato di mettere al centro dei miei interventi

si è manifestata anche nel corso di una riunione che abbiamo avuto poche settimane fa, insieme anche al coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, il prefetto Pecoraro, con il quale stiamo portando avanti una serie di iniziative per rendere più agevole l'individuazione dei responsabili di manifestazioni antisemite, ma che, in generale, si allargano allargano alla dimensione della mancanza di rispetto nei confronti degli altri. A ciò andrà aggiunto un efficace e tempestivo controllo sul rispetto rigoroso di tale assegnazione, prevedendo sanzioni nella misura in cui la società responsabile non si adoperi adeguatamente affinché, durante tutto lo svolgimento della partita, gli spettatori mantengono il posto assegnato. È nostra intenzione prevedere che le sanzioni comminate alle società sportive per gli episodi di antisemitismo e razzismo che avvengono in occasione delle manifestazioni sportive siano valide anche nei campionati successivi, con particolare attenzione anche all'inasprimento della pena in caso di recidiva. È stato avviato il percorso di approfondimento con il Garante della *privacy* per utilizzare sempre più intensamente la tecnologia per la sicurezza degli stadi e raggiungere l'obiettivo di responsabilizzare chi entra un impianto sportivo. Spero di poter portare gli esiti e gli approfondimenti in quest'Aula a stretto giro. È indubbio, infatti, che la necessità di stigmatizzare tali condotte, ritenute ingiustificabili e intollerabili, con determinazione, costanza e fermezza, deve consentire un intervento tempestivo che blocchi questi gesti offensivi, discriminatori e violenti, per non compromettere l'importante funzione educativa che lo sport fondato su valori etici universali ricopre nei percorsi di crescita, soprattutto dei più giovani. Un altro impegno concreto è quello di rivolgermi - come sto già facendo - alla Federazione italiana gioco calcio, alla Lega Serie A e B e alla Lega Pro, affinché si intervenga, in maniera decisa e sistematica, per coinvolgere i *club*, i tecnici, i calciatori, gli arbitri e tutti gli operatori del settore, nel promuovere, durante la stagione calcistica, campagne di sensibilizzazione contro l'odio e la discriminazione per motivi religiosi o razziali, nonché nel favorire un linguaggio inclusivo e libero da ogni pregiudizio e stereotipo. Ognuno nel proprio ruolo deve porre in essere le migliori azioni per garantire lo spettacolo sportivo e impedire che l'immagine del calcio italiano e dell'Italia intera siano compromessi da gesti del genere. Ritengo sia necessario, altresì, chiedere uno sforzo collaborativo e collettivo, perché si prevedano, nei regolamenti interni, norme rigide da applicare in modo univoco ogni qualvolta si verifichino gesti di razzismo negli stadi. Durante la presentazione dell'ottava edizione del rapporto dell'Associazione italiana calciatori «Calciatori sottotiro» è emerso un dato molto preoccupante e allarmante: la serie A è il campionato nel quale avvengono più episodi di minacce o intimidazioni contro i calciatori. È stato avviato lo scorso 31 marzo un tavolo congiunto con il ministro Piantedosi, al quale ho fatto riferimento nella mia introduzione, al quale hanno partecipato oltre che il Capo della polizia, il coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, il Capo della pubblica sicurezza, il Presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Presidente della Comunità ebraica di Roma, la Federazione italiana gioco calcio, la Lega serie A. Nel corso della seduta sono stati analizzati i recenti episodi avvenuti negli stadi ed è stata condivisa la presentazione di un documento del Governo per una maggiore responsabilizzazione del mondo del calcio anche attraverso il rafforzamento dello strumento del codice etico e l'implementazione di sistemi di videosorveglianza all'interno degli impianti. degli impianti. L'obiettivo è realizzare più efficaci azioni sia sul fronte del contrasto al grave fenomeno, perseguendo tempestivamente i responsabili di tali atti, sia su quello della prevenzione, con la partecipazione attiva degli stessi *club* calcistici e agendo, in particolare, sulle frange estreme delle tifoserie. L'impegno deve essere comune e il messaggio deve essere chiaro. Questo è un tema soprattutto culturale, che ha bisogno di strategie anche di lungo periodo, colpendo nell'immediatezza ma anche coinvolgendo in azioni mirate e complete la scuola, gli istituti accademici, le agenzie educative e le autorità governative che a vario titolo si occupano in particolare di formazione e di progettazione di percorsi educativi e di crescita.

Peraltro, sapevamo che c'era già in atto un importante lavoro da parte sua. Oggi lo ha confermato attraverso un vero lavoro di squadra - per rimanere nel linguaggio sportivo - perché bisogna coinvolgere tutti i protagonisti dello sport, in questo caso del calcio Il calcio è uno sport bellissimo, ma - come ha detto lei - la parola rispetto per noi è fondamentale, perché racchiude davvero tutti i significati. Ma quel rispetto noi lo chiediamo anche da parte dei *media*, perché l'informazione sia davvero plurale, attenta a stigmatizzare certi gesti e a responsabilizzare in maniera seria sia le società sportive, sia gli sia gli atleti, perché gli atleti - i calciatori in questo caso - sono i testimoni positivi a cui guardano i giovani, i bambini. Se vogliamo riportare i nostri ragazzi negli stadi e quindi costruire un modello diverso aperto alle famiglie, come già avviene in alcuni stadi, soprattutto in quelli che sono magari di proprietà della società come nel caso della Juve, ma anche di altre squadre, dobbiamo fare questo lavoro e debellare il fenomeno orribile di violenza e razzismo che purtroppo vediamo soprattutto nei livelli più alti, a cominciare dalla serie A. Concludo,

L'Italia potrebbe davvero diventare un modello nuovo con percorsi educativi di coinvolgimento nelle scuole, con un linguaggio più consono, e abbattere ancora quei muri di ignoranza che purtroppo vediamo ormai a tutti i livelli. Grazie, signor Ministro, e buon lavoro.

*(LSP-PSd'Az)*. Egregio Ministro, il Piano nazionale di ripresa e resilienza individua nello sport uno strumento importante di inclusione e coesione sociale, tanto più in contesti urbani dove esistono situazioni di grave disagio giovanile, e per questo destina risorse per interventi di costruzione e riqualificazione di impianti sportivi attraverso appositi bandi a favore dei Comuni. Con particolare riferimento a uno degli strumenti più efficaci delle politiche pubbliche governative in tema di sport, ossia il bando «Sport e periferie», è stato segnalato da più parti che i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11, risultano però troppo stringenti. Infatti numerosi soggetti beneficiari (Comuni di piccole dimensioni siti in zone a forte disagio socio-economico) hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni. Le motivazioni di tali ritardi sono riconducibili al costante stato di emergenza che si prolunga, per varie cause, ormai dal febbraio 2020. In particolare, la crisi energetica e dei prezzi delle materie prime dovuta principalmente alla guerra in Ucraina ha costretto i beneficiari ad apportare numerosi varianti ai loro progetti, al fine di poter realisticamente aggiudicare

la prossima scadenza delle concessioni degli impianti impedisca di fatto ai soggetti che ne gestiscono le attività di poter accedere a linee di finanziamento strumentali e a investimenti mirati nel rilancio delle strutture. Considerato che, Ministro, in sede di esame in Senato del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti - il cosiddetto decreto PNRR - è stato accolto l'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio, si chiede, quindi, a lei e al Governo quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo con riferimento ai suddetti interventi destinati al settore sportivo, al fine di garantire ai Comuni una utile e congrua flessibilità nella realizzazione di importanti progetti d'impiantistica sportiva, volti a incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, nel rispetto degli obiettivi del PNRR, anche mediante il rafforzamento e la stabilizzazione del sistema di garanzia alle linee di finanziamento per i soggetti gestori degli stessi impianti.

Signor Presidente, ringrazio il senatore Marti, che sa con quanta attenzione seguiamo questo tema, che coinvolge una pluralità di soggetti rispetto agli strumenti assegnati, e la ringrazio anche per aver fatto riferimento all'accoglimento dell'ordine del giorno G/564/28/5 (testo 2), che testimonia, appunto, la volontà di intervenire in tal senso con una probabilità di strumenti che non siano soltanto i singoli elementi. Entro nel merito delle questioni esposte per quanto riguarda in particolare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è stato assegnato al Dipartimento per lo sport con gli investimenti che sapete: 700 milioni di euro - permettetemi di lasciare agli atti anche un dato che ci fa riflettere - obbligatoriamente con 350 milioni per nuove edificazioni e consumo di territorio. Questo abbiamo trovato e con questo abbiamo lavorato attraverso tre linee di intervento. In adesione agli avvisi pubblicati in data 22 marzo 2023, relativi ai *cluster* 1, 2 e 3, all'esito della fase istruttoria, il Dipartimento ha ammesso al finanziamento 298 interventi. La *milestone* e *target* M5C2-21 ha fissato al 31 marzo 2023 il termine indicativo per l'adozione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla aggiudicazione degli appalti da parte dei Comuni soggetti attuatori. Ricordo che il cancello più delicato nonché il principale è quello del giugno 2026 per l'ultimazione dei lavori, la rendicontazione, la certificazione e quant'altro. Stiamo cercando di avere anche un via libera a fare in modo che il cancello del 31 marzo, appunto, venga rispettato nella sua indicatività rispetto alle perentorietà del dato, e su questo daremo evidenza. Quanto al *target* iniziale fissato per la notifica dell'avvenuta aggiudicazione di tutti gli appalti, alla data odierna risultano aggiudicate gare per 245 su 298 interventi; tra queste, le gare aggiudicate entro il 31 marzo 2023 si riferiscono a complessivi 241 interventi. I dati raccolti dimostrano il raggiungimento sia della *milestone* europea e nazionale di marzo 2023 per l'aggiudicazione delle gare d'appalto sia un cauto ottimismo per il raggiungimento del *target* di giugno 2026, che poi è quello principale, che prevede, come ho detto, il completamento di almeno 100 interventi, per una superficie complessiva di almeno 200.000 metri quadri. In relazione al bando «Sport e periferie», è già pronta la bozza del nuovo decreto di individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2023, ai fini della gestione del fondo, e la sua immediata pubblicazione con l'avviso «Sport e periferie 2023», per finanziare progetti fino a 75 milioni di euro, al quale potranno partecipare, anche qui, i Comuni ad oggi definanziati che non hanno potuto assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022. Questa mi sembra una prima risposta, con una misura immediatamente disponibile che ha caratteristiche pressoché equivalenti. Cercheremo nei criteri di dare priorità a quei Comuni che non hanno potuto beneficiare della continuità dei finanziamenti previsti e che quindi hanno la precedenza rispetto a quelli che si presentano per la prima volta. Mi preme evidenziare che nella legge di bilancio, approvata a dicembre, è stata inserita una norma per l'incremento dei fondi «Sport e periferie» di 50 milioni di euro dal 2023 al 2026. Credo che questo sia altrettanto importante per avere la certezza della continuità delle misure finanziarie. A ciò si aggiunga che la disposizione poi confluita nell'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, cosiddetto decreto PNRR 3, 3, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione provveda all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, che siano inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori, ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Tale disposizione è frutto anche dell'attività di questo Governo. In ultimo, al fine di favorire la realizzazione dei progetti di impiantistica sportiva, in particolare quelli rivolti a incrementare l'inclusione e l'integrazione sociale, stiamo supportando anche le prerogative dell'Istituto per il credito sportivo, che è un altro strumento di grande attualità e utilità, che con gli strumenti a sua disposizione fornisce fornisce un concreto e significativo ausilio nel perseguimento dei predetti obiettivi. Mi riferisco in particolare alla fornitura di forme di finanziamento a tasso zero, grazie ai bandi predisposti in collaborazione con l'ANCI, quali in particolare «Sport missione comune» e «Comuni in pista», ai quali si aggiunge «Sport verde comune», la nuova misura dedicata agli interventi di efficientamento energetico, e al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, che ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture e attrezzature sportive, comprese le relative aree, fino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso e con costi particolarmente contenuti, anche in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

e come lei stia tentando di muoversi, attraverso il Ministero, in questa insidiosa situazione. di mantenere dritta la barra che sta portando avanti da un po' di tempo, tentare di aiutare queste piccole comunità e i nostri amministratori a superare agevolmente questo problema, come tanti altri, perché per noi la scuola e lo sport sono al centro della ripresa e vanno aiutati. Quindi, grazie Ministro, anche a nome dei colleghi.

secondarie e strumentali delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche, quali attività derivanti da rapporti di sponsorizzazione o promozioni pubblicitarie, cessione di diritti, gestione di impianti e strutture sportive, nonché indennità legate alla formazione degli atleti; considerato che tale provvedimento, operante un vero e proprio riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, è entrato in vigore il 17 novembre 2022 e le misure relative invece al lavoro sportivo si sarebbero dovute applicare a partire dal 1° gennaio 2023; termine quest'ultimo spostato al 1° luglio prossimo

quindi chiederle cortesemente di sapere se il primo luglio 2023 sarà la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo o se siano prevedibili ulteriori proroghe e quali saranno i benefici per il mondo sportivo, complessivamente considerato.

quello della riforma dello sport, in particolare del lavoro sportivo. Rispondo già in estrema sintesi che, così come ho già avuto modo di anticipare in altri miei interventi, la data del primo luglio sarà quella di entrata in vigore della riforma, quindi mi auguro che ormai questo si sia già stabilizzato nei convincimenti di tutti, nell'interesse dell'intero sistema e soprattutto dei soggetti che fino ad oggi non hanno avuto tutele.

rispetto a ciò che avevamo trovato e che evidentemente aveva bisogno di ulteriori rifiniture, tenendo conto anche di quanto ci è stato messo a disposizione nel confronto con i portatori di interesse. Do al Senato un'informazione:

Non accetterei pertanto rinvii all'applicazione della nuova disciplina in tema di lavoro sportivo, perché non è immaginabile rimandare il doveroso riconoscimento della giusta dignità economica e finanziaria a chi lavora nel mondo dello sport e ne trae il sostentamento per sé e la propria famiglia: hanno diritto, come tutti gli altri lavoratori, a essere tutelate dagli enti previdenziali e assicurativi, sia sotto il profilo previdenziale sia sotto quello assicurativo, a ricevere tutela in tema di maternità, degenza ospedaliera, malattie, eccetera. Sinora la qualifica di soggetti non lavoratori, in quanto percettori di redditi qualificati come diversi dal legislatore tributario, ha determinato assenza di tutele, difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori e comportato inaccettabili differenze di trattamento che un Paese civile non può tollerare. Numerosi sono gli altri benefici per l'intero mondo sportivo: innanzitutto l'introduzione di una chiara disciplina sostanziale nel dilettantismo, la cui mancanza (quasi tutto è stato finora rimesso al legislatore tributario) ha determinato e continua a determinare difficoltà operative e forti incertezze interpretative, con il sorgere di numerosi contenziosi. Queste incertezze verranno risolte grazie ai criteri introdotti con la riforma del lavoro sportivo, che sono funzionali a mettere l'operatore in condizione di operare una corretta qualificazione e individuazione della figura del lavoratore sportivo e quindi a non incorrere nelle sanzioni per il caso di errato inquadramento che, per il loro ammontare, possono mettere in crisi la aziendale delle realtà sportive. Penso, ancora, alle misure di carattere fiscale ed economico finalizzate ad alleggerire enti e associazioni. Mi riferisco a misure come l'esenzione da tassazione fino a 15.000 euro di compenso; alla riduzione del 50 per cento fino al 31 dicembre 2027 della base imponibile per il calcolo contributivo; alla modifica del trattamento dei premi per evitare che questi siano ancora considerati, come avviene oggi, parte del compenso dell'atleta o del tecnico; alle semplificazioni da attuare attraverso il registro L'obiettivo è ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport e consentire in tal modo un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società dilettantistiche mediante l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche detenuto presso il Dipartimento per lo sport, che consentirà, non solo di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha effettivamente diritto, ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale.

Signor Ministro, mi dichiaro assolutamente soddisfatto della sua risposta per chiarezza, puntualità e completezza.

quel mondo e che incredibilmente, come ha detto lei, non erano state mai ascoltate. Questo, tuttavia, si incastona perfettamente nella visione del Governo, del nostro presidente Meloni, che ha voluto dare riconoscimento con un Ministero allo straordinario mondo italiano dello sport, operando una scelta di competenza, che è quella della sua storia, per la quale esprimo un profondo apprezzamento. Credo che ci siano le migliori condizioni per valorizzare questa rappresentanza dell'Italia, che è quella della nostra società migliore. che con quello che lei già sta ponendo in essere presso il Ministero e con il riconoscimento in Costituzione tra qualche mese dell'attività sportiva in ogni sua forma, ci sarà la possibilità di dare una vera tutela a un mondo che la merita, che l'aspetta da anni e verso il quale Fratelli d'Italia si sentiva obbligato, perché sempre nelle nostre previsioni programmatiche c'è stata questa intenzione. Siamo convinti dunque che non sia un caso che sotto la guida del Ministero da parte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

recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech"